del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368,

signor sottosegretario Fazio, siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un momento molto importante per la vita democratica del nostro Paese. Stiamo vivendo un momento storico; altri Paesi prima di noi sono passati in momenti simili, spinti dalla storia, incalzati da vicende umane drammatiche che avevano sollecitato le coscienze e interrogato l'opinione pubblica. Davanti a un vuoto legislativo si è sentita in molti altri Paesi del mondo l'esigenza di introdurre regole che andassero incontro ai problemi reali della vita delle persone. I primi ad avviare questo processo sono stati gli Stati Uniti, seguiti da molti altri Paesi, come ci ha ricordato molto bene il professor Veronesi ieri nel suo intervento. Nel nostro Paese è innegabile vi sia stata una accelerazione emotiva nell'*iter* di una legge di cui il Senato si stava già occupando per la drammatica vicenda di Eluana Englaro. Non trovo nulla di strano in questa accelerazione, anche se ritengo che avremmo bisogno di un clima diverso per lavorare e di un tempo adeguato per i necessari approfondimenti; trovo però un'anomalia il fatto che, sull'onda emotiva di una vicenda grave ma personale, il Senato voti una legge profondamente sbagliata, che va contro la Costituzione, contro la libertà degli individui e, signora Presidente, in controtendenza con le legislazioni di tutti i Paesi europei e di tutti i Paesi del mondo. Facciamo un passo indietro. Il motivo per cui si è sentita l'esigenza di una legge sulle direttive anticipate di volontà è semplice: la Costituzione sancisce un diritto in base al quale nessun individuo può essere sottoposto ad una terapia contro la sua volontà. Questo diritto non è tuttavia applicato alle persone che hanno perso la capacità di intendere e di volere e con essa quella di esprimersi e di dare il proprio consenso alle terapie. Il motivo, signora Presidente, è molto semplice: i nostri Padri costituenti, scrivendo anche quel mirabile articolo 32 della Costituzione, hanno tenuto conto del momento storico e scientifico in cui vivevano; vivevano nel 1947. Il primo respiratore automatico è stato inventato nel 1952, la prima nutrizione artificiale alla fine degli anni '60: non non potevano immaginare che da lì a pochi anni ci sarebbe stata la possibilità di mantenere artificialmente in vita una persona che, però, non poteva più verbalmente esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso alle terapie. Ci si è posti dunque il problema di garantire tale diritto a tutti, guidati dal principio secondo cui la perdita della coscienza non si possa tradurre in perdita dei diritti. Assieme a 101 senatori avevo proposto un disegno di legge di cui non si è tenuto conto nella maniera più assoluta. Quel progetto si proponeva due obiettivi davvero semplici: il primo era scongiurare il rischio dell'accanimento terapeutico, garantendo a tutti la possibilità di lasciare indicazioni sulle terapie considerate accettabili e quelle non accettabili, se un giorno ci si trovasse nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso;

Purtroppo questa legge non risponde a nessuno dei due obiettivi sopra citati. Ciò significa che, se entrerà in vigore, un paziente ricoverato in una rianimazione con un tumore in fase terminale, con metastasi al cervello, sottoposto alla dialisi, a trasfusioni di sangue e alla nutrizione artificiale, non potrà essere accompagnato al momento più imperscrutabile della sua vita con la semplice sospensione di tutte le terapie, ormai utili solo a prolungarne l'agonia. Il medico non potrà chiamare la famiglia e chiedere quale fosse l'orientamento del paziente, quali le sue volontà e prendere in questo modo, in maniera umana, collegiale e trasparente, la decisione se interrompere o meno tutte le terapie ormai divenute futili. Forse quel medico, secondo la sua preparazione e il suo buon senso, interromperà lo stesso quell'inutile agonia, ma lo farà da solo, in silenzio, senza documentare l'interruzione di tutte le terapie nella cartella clinica. E questo non è quello che vorrei vedere accadere nel mio Paese. Con la legge che si vuole votare, se una persona lascerà un testamento biologico, il medico non sarà nemmeno tenuto a rispettare quelle volontà: fatto che mi sembra sufficiente per far sì che nessuno scriva mai un documento, sapendo che nel momento cruciale non sarà tenuto in considerazione. Sul secondo aspetto, l'introduzione del capitolo sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, mi pare vi sia da parte della maggioranza un atteggiamento di totale disattenzione ai più deboli. Il relatore ci ha ricordato che esiste un accordo con la Camera dei deputati, che sta lavorando ad un testo di legge sulle cure palliative. Per questo motivo una serie di emendamenti presentati in Commissione sanità dall'opposizione sono stati considerati inammissibili. Sinceramente, mi domando se i cittadini italiani, per cui noi lavoriamo, siano in grado di capire una tale giustificazione e se siano d'accordo sul fatto che un'intesa informale tra i due rami del Parlamento sia più importante di una risposta concreta ai loro problemi oggi, non domani. È vero che la Camera sta lavorando sulla questione, ma noi conosciamo bene quali siano i tempi e gli ostacoli che si possono incontrare nel corso dell'*iter* di una legge. Intanto, però, la Lombardia ha 38 *hospice* e la Sicilia, con 5 milioni di abitanti, soltanto 3. Senatrici e senatori, vi chiedo di dare un segnale al Paese, alle persone in maggiore difficoltà e almeno di inserire nella legge una norma sulla possibilità di prepensionamento per uno dei due coniugi nel caso in una famiglia vi sia la necessità di assistere un disabile grave o gravissimo, come un figlio o una figlia in stato vegetativo persistente. Infine aggiungo due ultime considerazioni. L'articolo 3 della legge si occupa dell'idratazione e della nutrizione artificiale, che non possono essere oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nella formulazione attuale, tali disposizioni si applicano soltanto ai soggetti in stato vegetativo, cioè a meno di 3.000 persone in tutto il Paese. Ma davvero stiamo facendo tutto questo per una legge che riguarderà lo 0,005 per cento della nostra popolazione? Non voglio dire che siano persone meno importanti, tutt'altro, ma non dovremmo porci il problema anche di tutti gli altri? Che risposte diamo alle centinaia di migliaia cittadini che ogni anno vivono senza tutele le fasi finali della loro esistenza? Faccio queste affermazioni perché sia chiaro a tutti che la maggioranza non vuole fare una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento: vuole fare una legge per impedire l'esercizio della libertà ad alcuni individui sulle questioni che riguardano la fine della loro vita, perché questa legge impone ai cittadini una scelta morale, decide per loro, privandoli di un diritto fondamentale. La scelta di continuare o di sospendere le terapie, e di accettarne le conseguenze, è una questione morale, sarete d'accordo con me. La legge di uno Stato laico e democratico non deve occuparsi delle scelte morali, ma delle scelte giuridiche, all'interno delle quali la scelta morale possa essere liberamente esercitata da ciascun cittadino. Io vi chiedo di non approvare questo testo così come è uscito dalla Commissione sanità, perché con esso il Paese andrà incontro a problemi più complessi di quelli attuali: si andrà incontro ad una lacerazione politica profonda, i cittadini si rivolgeranno ai tribunali per vedere rispettati i propri diritti, i medici si troveranno nell'imbarazzante situazione di dover scegliere se trasgredire la legge per tenere fede all'alleanza con i pazienti, che io considero sacra, oppure a venire meno al loro codice deontologico. Vogliamo davvero tutto questo? Signor Presidente, fermiamoci a riflettere ancora. finestra"). La senatrice Franca Chiaromonte, iscritta a parlare in discussione generale e presente in Aula, deposita il testo scritto del proprio intervento. Grazie, senatrice Chiaromonte. Presidente, Governo onorevoli colleghi, la presentazione nelle ultime tre legislature di numerosi disegni di legge in materia di dichiarazioni di volontà anticipate per i trattamenti sanitari è è stata indice della consapevolezza, anche in ambito parlamentare, della necessità di un intervento normativo in materia. Su questo delicatissimo argomento il passato Governo di centrosinistra ha usato i suoi due anni per svolgere audizioni senza però mai attivare e avviare discussioni che portassero alla predisposizione di provvedimenti concreti. Per questo Governo, invece, questo disegno di legge è stato fra i primi provvedimenti incardinati a partire dal mese di ottobre. Certo, il caso Englaro ha accelerato i tempi ma noi comunque abbiamo sempre creduto nell'indispensabilità di una regolamentazione sul tema del fine vita. vita. A questo proposito in Parlamento la discussione e il dibattito sono stati serrati, ma con posizioni politiche generali chiare. Abbiamo in Parlamento una maggioranza - questa maggioranza che vuole la legge, anche se si divide nella discussione su come articolarla, ed un'opposizione che, invece, non vorrebbe nessuna legge o per un estrema radicalizzazione o per un fondamentalismo di carattere religioso. Che la legge sia necessaria, però, è confermato da una serie di posizioni e di eventi; posizioni ed eventi laici, laddove anche la scienza, nonostante i continui progressi, non ha ancora alcuna certezza su questo tema, e posizioni ed eventi religiosi con gli interventi sull'argomento, tra gli altri, anche di pontefici come papa Paolo VI nel 1970 e papa Benedetto XVI nell'Angelus della domenica *in albis* dell'anno scorso. Noi oggi stiamo cercando di fare una legge che sia la più equilibrata possibile, la più condivisa possibile perché crediamo che, dopo tanti anni, si debba passare finalmente dalle parole ai fatti, coniugando il diritto alla vita con la libertà di cura e dicendo però no all'eutanasia di Stato, da un lato, e all'accanimento terapeutico dall'altro. Certo, sull'idratazione e sull'alimentazione i pareri non sono omogenei, ma sicuramente siamo molto meno divisi di quel che appare in quest'Aula. Per ora io fra tanti, ma veramente tanti dubbi, ho una sola certezza: una persona, se deve morire perché malata irrimediabilmente, non continua a vivere solo perché le si introducono dei liquidi attraverso una vena o un sondino; se invece chiudendo quell'unica somministrazione muore, io faccio dipendere quell'effetto dall'avere interrotto un atto basilare di aiuto alla vita indispensabile. Ciò premesso, ribadisco, come già ho fatto in Commissione giustizia relazionando sul parere al disegno di legge, che il testo unificato intende riaffermare, nel pieno rispetto del diritto positivo e *in primis* della Costituzione italiana, il valore involabile della indisponibilità della vita. E sottolineo come con il medesimo si sia tra l'altro data immediata e puntuale esecuzione alla mozione recentemente approvata dal Senato, con cui si auspicava l'urgente approvazione di norme che garantissero la certezza di cure idonee e di adeguata assistenza nella fase terminale dell'esistenza, ovvero quando le condizioni personali non consentissero di provvedere in maniera autonoma alle necessità vitali fondamentali, nella piena convinzione che in Italia nessuno debba più morire di fame e di sete. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, credo sia giusto ricordare, anche se è stato già fatto, che la questione del cosiddetto testamento biologico e delle tematiche ad esso collegate non è di oggi. Essa è infatti all'ordine del giorno del dibattito politico da trent'anni, da quando nel 1976 il caso Quinlan, come ha ricordato lo stesso professor Veronesi, scosse l'opinione pubblica statunitense e poi rimbalzò in tutti i Paesi avanzati, dove i crescenti progressi delle conoscenze tecnico-scientifiche avevano già prodotto interrogativi tali da mettere a soqquadro le convinzioni e dilaniare le coscienze. Questa notazione è la dimostrazione di quanto laceranti, difficili, drammatici per la coscienza di ciascuno e al di là degli schieramenti di parte, siano gli argomenti che come questo aprono problemi etici di complessità incredibile. Non è davvero un caso, credo, che tre decenni non siano bastati ai legislatori che si sono succeduti in questa e nell'altra Aula del nostro Parlamento per iscrivere la materia in un quadro di regole certe e condivise, perché molto semplicemente si tratta di una materia difficile, di una materia delicata che, complice il processo ipertecnologico di crescita della nostra medicina, apre dilemmi fin qui estranei al percorso umano. Credo di esprimere un pensiero in quest'Aula largamente condiviso se affermo che l'accelerazione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame sia stato prodotto dalla controversa e drammatica conclusione del caso Englaro, che ha trovato la risposta ai dilemmi, agli interrogativi, alle istanze, alle richieste che prima ricordavo in una sentenza della magistratura; laddove questa è intervenuta evidenziando che non poteva farsi diversamente, atteso che vi era un *vulnus* legislativo, al quale peraltro la magistratura stessa chiedeva di porre rimedio. Un fatto grave, questo, che non sia l'organo sovrano espressione della volontà popolare a dare un'indicazione e una risposta, ma sia un altro potere costituito della nostra democrazia. Questo riferimento è utile ad inquadrare la cornice di oggettiva difficoltà dentro la quale dobbiamo provare a ragionare (e sottolineo provare a ragionare), rifuggendo dalle tentazioni di radicalizzare il confronto e di ingessarlo nei presunti dogmatismi di opposte e non conciliabili verità. Sono sempre stato convinto fin dall'inizio dei lavori in Commissione sul testo del senatore Calabrò (al quale voglio indirizzare in questa sede, una volta di più e con grande affetto un pubblico attestato di stima e un sincero ringraziamento per l'onestà intellettuale l'umiltà tenace con la quale ha portato avanti questo provvedimento), che il punto centrale della delicatissima questione che ancora discutiamo sia tutto nella risposta ad un'unica domanda: fino a che punto la vita di una persona può essere considerata un Un interrogativo che è andato ben oltre l'iniziale tema che lo aveva generato, caro collega Marino, relativo al fatto se l'alimentazione e l'idratazione fossero sostentamento vitale o trattamento sanitario e come tale dunque configurabile come accanimento terapeutico. È infatti sulla vita come bene disponibile che si registra la divaricazione tra chi ritiene che ciascuno, in nome del sacro ed inviolabile principio di libertà, possa fare della sua vita ciò che più e meglio ritiene e chi al contrario ritiene che la libertà assoluta di disporre di sé sia costitutivamente in antitesi con i princìpi e le regole del vivere civile e sociale e quindi non ammissibile. Come è evidente, si tratta di posizioni inconciliabili, espressioni di concezioni, sensibilità e culture profondamente diverse dei valori fondanti dell'esistenza. Dirò subito, per chiarezza, che sono tra coloro che ritengono che la vita sia un bene indisponibile e non negoziabile. Aggiungerò anche che avverto un po' di disagio quando, anziché confrontarci su argomenti opponendo posizione a posizione, vi è chi considera pregiudizialmente la mia convinzione come frutto di un dogmatismo confessionale e fideistico. A ben vedere, è proprio questo l'atteggiamento che rende più difficile il dialogo: il rifiuto di molti a prendere in considerazione, con la serenità che sarebbe invece necessaria, il fatto che il principio della indisponibilità della vita non è sostenuto solo da argomenti teologico-confessionali, ma anche da forti e ben radicati argomenti laico-razionali. Vi è chi come il professor Francesco D'Agostino, presidente onorario del Comitato nazionale per la bioetica (ma vi sono accanto a lui illustri Presidenti emeriti della Corte costituzionale), si è speso molto per affermare questa verità, spiegando - direi autorevolmente come quello della indisponibilità della vita sia con buona pace dei laicisti un principio aristotelico ancor prima che cristiano, ricordandoci che la stessa verità è stata poi variamente ribadita da giganti del pensiero della statura di Kant o di Schopenhauer (sì, anche lui, il nichilista Schopenhauer!), entrambi concordi nell'affermare che la vita non è bene di cui il singolo possa disporre a suo piacimento, anche se sulla base di considerazioni del tutto diverse e per non dire singolarmente opposte. È però all'Aristotele dell'Etica Nicomachea che bisogna riferirsi per significare come il concetto della indisponibilità della vita sia assolutamente precristiano. Il filosofo argomentava contro il suicidio, sostenendo che l'individuo appartiene alla *polis* e non ha dunque il diritto di privarla della sua presenza e della sua attività. Il professor D'Agostino non parla ovviamente né di *polis* né di Patria, né di Stato, ma osserva che ognuno di noi vive all'interno di una rete di relazioni interpersonali. Quindi, sostiene il bioeticista - che cito alla lettera - «chi ritiene di avere il diritto di poter disporre della propria vita arriva di fatto a disporre - magari senza rendersene conto - di tutta la rete di relazioni interpersonali (che sono familiari, amicali, lavorative, politiche, sociali), al cui interno si è formato come persona e che hanno contribuito a costituire e costruire la sua identità. Uscendo da questo mondo e ritenendo di averne il diritto, egli si comporta ingiustamente con tutti coloro che hanno interagito nel passato e che potrebbero in futuro ancora interagire con lui, che cioè hanno messo, o comunque potrebbero aver messo a disposizione sua il proprio patrimonio di esperienze». In questa interdipendenza di individui, che l'elemento irrinunciabile e fondante dell'esperienza umana e della stessa idea di società, risiede dunque il nocciolo della questione. Non apparteniamo solo a noi stessi ma anche alla rete di relazioni interpersonali che ha fatto e fa di noi quel che siamo. Ritenere disponibile dunque la vita umana significa infliggere un *vulnus* fatale alla possibilità stessa della dimensione sociale, per la quale la vita non è soltanto un valore accanto accanto ad altri valori ma è il presupposto della stessa elaborazione sociale di ogni valore. Ecco perché il principio dell'indisponibilità della vita non è negoziabile, perché se lo discutessimo mineremmo le pietre d'angolo su cui appoggiano le fondamenta del nostro modello di civiltà, con conseguenze incalcolabili per il futuro. E a tutti coloro che arrivando talvolta a promuovere, sotto le spoglie suadenti della *pietas,* la causa del diritto a disporre della propria esistenza, aprendo così la porta ad una deriva nichilista, gioverà ricordare che se questa civiltà, della quale siamo al tempo stesso eredi e artefici, è stata possibile è esclusivamente sulla base dell'affermazione di questo principio: se avesse prevalso, al contrario, il concetto della vita come bene disponibile, forse saremmo ancora dalle parti della rupe Tarpea. Su questo punto fondamentale non mi è sembrato di registrare, a meno di colpevoli distrazioni, controargomentazioni convincenti condotte in punta di ragionamento; eppure, torno a dirlo, proprio su questo punto nodale dell'intera questione si svolge il ragionamento. Se infatti attraverso un confronto aperto, sereno arrivassimo a condividere la convinzione, tutta laica, razionale e soprattutto fondata sull'irrinunciabile dimensione sociale del nostro essere persone, in ordine all'indisponibilità della vita, credo che al provvedimento che oggi stiamo discutendo in Aula si aprirebbe una strada in discesa. Il lavoro in Commissione ha dato ampia prova del fatto che esistono margini per arrivare ad una legge formulata con il contributo, anche necessario, di culture e sensibilità differenti. Lo ha ribadito il senatore Calabrò, con specifico riferimento ad alcuni aspetti critici che sono stati utilmente dibattuti, analizzati e migliorati, e lo ha confermato, con un'onestà intellettuale che è tutta da apprezzare, il senatore Gustavino, riconoscendo che il testo della legge è uscito dalla Commissione migliore di come vi era entrato. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente, chiedendo un ultimo minuto. Voglio coltivare l'auspicio che questa discussione generale, per questa volta e per questa specialissima occasione, si sottragga alle logiche dei discorsi fatti per lasciare traccia nei resoconti; che questa Aula torni ad essere, come siamo in tanti ad auspicare, come emerso nell'interessante dibattito sulle riforme che abbiamo svolto ieri, il luogo dove non solo si approvano le leggi ma dove si forma e si costruisce il pensiero che le origina. Eppure non può non prendersi atto delle oggettive difficoltà a trovare le necessarie convergenze, attese le dichiarazioni tanto amare quanto vere della vice presidente Bonino, quando afferma che a dividerci nella sostanza è una diversa lettura dell'articolo 32 della Costituzione. Ragionando ai bordi di questo solco, dunque, potrà forse anche essere vero che in democrazia mi rivolgo soprattutto alla illustre collega Bonino - i numeri non sempre coincidono con il diritto, ma è ancora più vero che dietro la forza dei numeri in questa occasione c'è anche la forza dei princìpi, dei valori, delle convinzioni e anche dei ragionamenti svolti con la massima apertura al confronto con le ragioni altrui. Non c'è una logica muscolare dietro e dentro il testo di questa legge, ma la traduzione, anche difficile e sofferta in alcuni momenti, di un lungo percorso di impegno, di riflessione e confronto. Questo ritengo giusto ricordarlo, con serenità, con pacatezza e con grande convinzione, assumendo la responsabilità, non solo etica, del mio sostegno alla legge*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, senatore relatore, onorevoli senatrici e senatori, lunedì 9 febbraio, durante i lavori del Senato sul disegno di legge sul caso Englaro, Eluana muore. In quel clima drammatico, dove alcuni irresponsabili colleghi della destra ci gridano "assassini", un barlume di ragione fa sì che qualcuno concordi con il Presidente del Senato che è meglio rinviare il voto sulle due mozioni presentate. Venerdì 6 febbraio, infatti, il Governo aveva stressato la Costituzione e il Paese adottando un decreto-legge, pur nella consapevolezza che il Capo dello Stato non lo avrebbe controfirmato. Nella stessa serata, il Governo ritira il decreto-legge trasformandolo in disegno di legge. Contestualmente, la maggioranza decide di lanciare una sfida al Parlamento e al Paese, dandosi l'obiettivo di approvare la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento in soli tre giorni. Inizia il mio personale calvario che, inevitabilmente, ha riflessi sulla sfera del mio ufficio di senatore della Repubblica. Il testo del disegno di legge viene diffuso ed è chiaramente articolato come una legge *ad personam* contenente, in questo caso, il principio della non negoziabilità del diritto alla vita. Quindi è un disegno di legge che serve ad ottenere almeno due obiettivi: intervenire in una situazione giuridica soggettiva sulla quale ha statuito una sentenza della magistratura passata in giudicato e interrompere con effetto immediato il protocollo di progressiva riduzione dell'idratazione e dell'alimentazione previsto nella sentenza relativa ad Eluana Englaro. Per noi senatori, quella sera del 9 febbraio, il disegno di legge significa, nei fatti, scegliere, essere obbligati a scegliere, tra il non fare nulla (e cioè rassegnarsi alla progressiva diminuzione dell'alimentazione e dell'idratazione di Eluana, di una persona umana, portandola alla cessazione della sua esistenza) e il permettere che Eluana continui a sopravvivere al proprio strazio. Siccome ogni spiegazione, ogni interpretazione,

Siccome ogni spiegazione, ogni interpretazione, è per definizione insufficiente a circoscrivere il perimetro del campo del quale avremmo dovuto occuparci con quel disegno di legge, il groviglio di inquietudine, coscienza, ricordi personali di situazioni simili già vissute nella mia vita (due volte, con due diverse soluzioni finali) fa di quel fine settimana, dal 6 febbraio al 9 febbraio, uno dei più bui e angosciosi della mia vita personale e di senatore. Eluana muore verso le ore 21 e in Aula il dibattito sul disegno di legge viene interrotto. Signora Presidente, nel dibattere sul disegno di legge posto oggi all'attenzione dell'Assemblea, il frutto più evidente della semplificazione è rappresentato dal conflitto tra due posizioni antitetiche, l'una assertrice dell'autodeterminazione del singolo e l'altra dell'inviolabilità della vita umana. La realtà che emerge dal disegno di legge proposto dalla maggioranza è assai diversa: riguarda solo indirettamente la libertà di rinunzia ai trattamenti medici, in quanto in qualsiasi momento il paziente o chi per lui può rinunciare al ricovero e così sarà anche con la legge Calabrò oggi in discussione. Il disegno di legge esclude, piuttosto, che il medico si renda compartecipe di una scelta del paziente che contrasti con il suo codice deontologico, il quale codice già oggi vieta i comportamenti indicati nel testo Calabrò. La posta in gioco è un'altra: essa riguarda il fatto se il medico si debba rendere compartecipe della decisione del paziente anche quando questa vada contro la propria deontologia, così da consacrare per legge gli esiti della vicenda Englaro. Ecco allora come appare una forzatura e una mistificazione quella che caricaturizza il paziente attaccato forzosamente al sondino. La medicina odierna dispone ormai di mezzi in grado di ritardare artificialmente la morte, senza che il paziente ne riceva un reale beneficio: lo ha detto ieri il senatore Veronesi. Il paziente viene semplicemente mantenuto in vita - o si riesce solo a protrargli di qualche tempo la vita - a prezzo di ulteriori e dure sofferenze. Si può determinare, in taluni di questi casi, il cosiddetto accanimento terapeutico, consistente nell'uso di mezzi particolarmente sfibranti e pesanti per il malato, condannandolo di fatto ad un'agonia prolungata artificialmente. L'alimentazione e l'idratazione, anche artificialmente amministrate, devono quindi rientrare tra le cure normali dovute sempre all'ammalato a patto che non risultino gravose per lui. Diversamente, la loro indebita sospensione può avere solo il significato di vera e propria eutanasia. Per il medico e i suoi collaboratori, allora, non si tratta di decidere della vita o della morte di un individuo. Si tratta semplicemente di essere medico, ossia di interrogarsi e decidere in scienza e coscienza quale cura rispettosa del vivere e morire sia utile e necessaria per l'ammalato a lui affidato. Questa responsabilità non esige il ricorso sempre e comunque ad ogni mezzo. Può anche richiedere di rinunciare a dei mezzi per una serena e, per alcuni di noi, cristiana accettazione della morte inerente alla vita. Può anche voler dire rispetto della volontà dell'ammalato che rifiutasse l'impiego di taluni mezzi nell'ambito di una decisione presa nel quadro sistemico che ho prima provato a tracciare. Colleghi senatori, stiamo parlando di complessità e non di chili di frutta da comprare al mercato. La complessità richiede ragionamenti approfonditi, distinguo e precisazioni. Ecco allora che mi spaventano quali non vedono l'ora di contarsi su posizioni radicali o dirompenti, nell'un senso o nell'altro. Parliamo della vita delle persone umane, della grazia ricevuta da un incredibile dono della natura, stiamo parlando di qualcosa molto più grande di noi che non è liquidabile con le mediazioni terminologiche che tranquillizzano le singole posizioni politiche, ma che non sortiscono alcun effetto sostanziale perché si perdono nel mare delle mediazioni del politichese. Condivido l'impegno nel difendere la necessità di legiferare su questa materia, ma non riesco ad approvare l'incitazione a ritenere giusto l'atroce epilogo della vicenda di Eluana Englaro. Come si può ritenere un diritto l'autodeterminare la propria vita, nel senso di respiro, calore, circolazione del sangue*,* pulsazioni, battito del cuore, insomma espressione di essere creatura vivente per un "volere" che non ci appartiene, in quanto originato da un misterioso evento naturale o sovrannaturale a cui la scienza, mi pare, abbia abbia finora fornito solo blande e parziali spiegazioni? Temo si stia affermando sull'argomento un sostanziale equivoco che vorrebbe avere nei concetti, rispettivamente, di vita e di vitalità lo stesso significato e che spiegherebbe il motivo per cui, a volte, di fronte a persone che hanno perso la vitalità, cioè la possibilità di muoversi, parlare, sorridere, cantare e ballare, si sia emotivamente portati ad affermare: se mi succedesse fatemi morire. Ma se una frazione di secondo prima di subire il trauma che determinerebbe lo stato in cui si è trovata Eluana ci si ravvedesse e si capisse che è comunque meglio vivere e si desiderasse improvvisamente il contrario? Ho sentito dire da un collega senatore che, per amore, in circostanze analoghe a quella di Eluana, si vorrebbe che per i propri amati figli si facesse la stessa scelta. Io non voglio nemmeno pensare di trovarmi in simili circostanze, ma provo a chiedermi se un familiare che ama con la stessa mia intensità preferirebbe piangere su una fredda tomba oppure tenersi il calore del proprio caro, a qualsiasi condizione, fino alla morte naturale e non a quella clinica. Non vi è dubbio che la prima è la più sbrigativa, ma io ringrazierò all'infinito mio padre, che ha scelto la seconda. Egli ha avuto ragione perché, pur nella difficoltà giornaliera imputabile agli anni della sua lunga e grave disabilità, oggi non potrei raccontare di aver vissuto in una grande e straordinaria famiglia, di essermi laureato, di avere una donna meravigliosa al mio fianco e tre figli favolosi, di essere stato quello che sono e di essermi impegnato fin da ragazzo nella politica e nello scoutismo cattolico, i cui valori inneggiano alla vita e non al diritto di morire. *(Applausi).* Come padre non capisco l'ostinata battaglia del signor Englaro, ma non mi permetto di giudicarlo; e mi rifiuto di unirmi a coloro che hanno visto in lui il desiderio di disfarsi di un "problema". La ragione naturale insegna che l'uomo, il medico (e chiunque abbia l'ufficio di assistere il suo prossimo), ha il diritto e il dovere, in caso di malattia grave, di adottare le cure necessarie per conservare la vita e la salute. Tale dovere - che egli ha verso se stesso e verso la società umana e, più spesso, verso determinate persone - deriva dalla giustizia sociale e anche dalla stretta giustizia, come dalla pietà verso la propria famiglia. Ma tale dovere non obbliga, generalmente, se non all'impiego dei mezzi ordinari (secondo le circostanze di persone, di luoghi, di tempo e di cultura), ossia di quei mezzi che non impongono un onere straordinario per se stessi o per altri. Un obbligo più severo sarebbe troppo pesante per la maggior parte degli uomini e renderebbe troppo difficile il raggiungimento di beni superiori e più importanti. I diritti e i doveri della famiglia dipendono, in generale, dalla volontà presunta dell'infermo incosciente, se egli è maggiorenne e *sui juris*. Quanto al dovere proprio e indipendente della famiglia, esso non obbliga, abitualmente, che all'impiego dei mezzi ordinari. se il tentativo di rianimazione costituisce per la famiglia un onere che in coscienza non si può ad essa imporre, questa può lecitamente insistere perché il medico interrompa i suoi tentativi, ed il medico può lecitamente acconsentire. Considerazioni d'ordine generale permettono di credere che la vita umana continui fino a che le sue funzioni vitali - a differenza della semplice vita degli organi - si manifestano spontaneamente o sia pure con l'aiuto di procedimenti artificiali. In gran numero di tali casi, essi formano l'oggetto di un dubbio insolubile e debbono essere trattati secondo quelle presunzioni di diritto e di fatto di cui abbiamo parlato. In conclusione, signor Presidente, cari colleghi, se battaglia in Parlamento ci deve essere, questa deve mirare a far sì che la gestione di tali drammatiche situazioni della vita non ricada esclusivamente sulla famiglia che le sopporta, le cui enormi difficoltà, di ogni genere, non possono essere rappresentate da qualche politico strillone ammantato di sacro furore ideologico.

senza poi assumersi l'onere di corrispondere la dovuta copertura finanziaria per passare dalle affermazioni di principio ai fatti, finendo così per confermare che non si vuole realizzare ciò che ad alta voce si sbandiera? Credo che questi siano temi difficili e complessi su cui è meglio non avere certezze, ma chiarezza del senso del limite. Non intendo avventurarmi, come altri hanno fatto, sul terreno di ciò che è morale e ciò che non lo è: va oltre il terreno del legislatore. Non amo vivere in uno Stato in cui siano i princìpi di una qualsiasi religione a impormi regole, ma ho anche timore di leggi dello Stato che possano costituire la premessa per decisioni che stabiliscano chi ha diritto di vivere ed avere assistenza e chi di morire senza riceverne. Grazie a tutti, veramente, per la pazienza. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci ritroviamo oggi in Aula a legiferare su un argomento così intimo e personale che fa parte della sfera di vita e familiare di ciascuno di noi, e che ha preso spunto da un fatto che ha coinvolto e sconvolto le coscienze di tutti, portandoci a riflettere, ormai da diversi mesi, su un tema essenziale sotto l'aspetto etico, umano e anche giuridico. Quindi, oggi ci troviamo, signora Presidente, a esaminare il testo pervenuto in Aula in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento. Un testo che è stato elaborato in maniera sofferta da tutti i colleghi della 12a Commissione, che noi ringraziamo per il lavoro svolto, da tutti, nessuno escluso. Questo perché su determinati temi le posizioni preconcette possono essere superate; infatti, molti ragionamenti sono stati motivati più da considerazioni personali che da contrapposizioni politiche. Il tutto con l'intento e l'obiettivo di rispettare la libertà e la persona per un verso, e sancire dall'altro l'inviolabilità della vita umana. Questo traspare appieno, è tangibile nel testo pervenuto in Aula, un testo che rappresenta un'efficace sintesi delle molteplici posizioni che si sono venute a trovare in campo. Un difficile compito questo, per il quale dobbiamo ringraziare il presidente della Commissione Tomassini, il relatore Calabrò e tutti gli altri. Dobbiamo però anche riconoscere i diversi tentativi di dare un contributo fattivo da parte della minoranza. Sul tema fondamentale, per noi intrattabile, dei trattamenti di alimentazione e idratazione artificiali, infatti, affermando che questi non costituiscono una terapia bensì forme di sostegno vitale, si possono creare le basi per convergenze su molte altre problematiche. L'attenzione e la cura poste nella chiarezza della stesura del testo sono poi indicative di una volontà comune di non lasciare adito ad errate interpretazioni, al fine di contenere ogni futura possibilità di equivoco e perché sia chiaro che alimentazione e idratazione artificiali non possono essere assimilate a forme di accanimento terapeutico e quindi non possono formare oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. In questo testo non sono previsti comportamenti assimilabili al suicidio assistito, come da qualcuno ventilato. È appunto sancito il diritto alla vita e alla sua indisponibilità proprio sulla stessa Carta costituzionale, incentrata su valori volti alla promozione e alla tutela della vita. Lo strumento del consenso informato diventa ora vincolante. Le disposizioni espresse dal soggetto nel testamento biologico diventano tali, come è giusto che sia. Ma non si afferma la propria volontà in modo presunto ed *ex post*. La volontà della persona deve essere certificata e non ricostruita. Dopo attente valutazioni con il medico, che recepisce la volontà dell'assistito, le DAT consentono invece la possibilità del rifiuto dei trattamenti sanitari da parte del paziente del paziente in vita, senza però stabilire per esso il diritto alla libertà di morire e comunque alla luce della tutela costituzionale del diritto alla salute, quale bene per la persona e per la società. Persino il documento del Comitato nazionale di bioetica del 2003 sottolineò il principio del *favor vitae* con un testo che vide concordi laici e cattolici. E proprio per questo le figure del medico di medicina generale (l'unico che possa fornire le giuste informazioni ai pazienti in virtù della professione esercitata e del giuramento d'Ippocrate)

Il paziente infatti da solo non può essere in grado di prendere decisioni così importanti e così specifiche, neanche quando è in condizioni di intendere e di volere, e diventano quindi figure determinanti soprattutto nel momento in cui si verifichi la possibilità di una volontà che per forza di cose non può essere espressa o aggiornata quindi motivata dai nuovi eventi, anche in relazione ai progressi della scienza medica e delle biotecnologie. Certamente il medico non può cagionare la morte del paziente o comunque non può recepire volontà in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica e professionale. Il caso Englaro ha scosso gli animi di tutti, ma ci ha resi sempre più convinti che lo Stato debba farsi carico di opportune iniziative volte ad aiutare e sostenere tutte le famiglie che vivono questi drammi, nel rispetto pieno delle competenze regionali in materia sanitaria, affinché esse non si sentano abbandonate dalla società civile e possano tutelare e assistere al meglio i loro congiunti. Nell'auspicio che tale provvedimento possa essere un esempio per misurare la maturità della nostra società e un condiviso comune punto di partenza per la certezza della vita e per la tutela dei diritti personali, signora Presidente, esprimo il mio plauso e la mia convinta adesione al testo pervenutoci oggi in Assemblea ed elaborato dalla Commissione sanità. Grazie Presidente, colleghi e colleghe, mi sia consentito, al principio del mio intervento, sottolineare la necessità di una legge sul testamento biologico, ma prima ancora quella della discussione su un tema come quello del fine vita. E perché essa testimoni la maturità della democrazia del nostro Paese, il confronto dovrebbe essere il più ampio possibile e il più possibile sottratto alla speculazione politica. Vicende dolorose come quella di Eluana Englaro e le migliaia di drammi analoghi che ogni giorno si consumano in silenzio nel nostro Paese, al di là dell'emotività istantanea, interpellano nel profondo le nostre coscienze e impongono al legislatore di dare una risposta certa, «non più procrastinabile», per cogliere il monito del Presidente della Repubblica. Nel definire indispensabile un intervento legislativo sul fine vita, il Capo dello Stato ha auspicato «il massimo sforzo di convergenza, in Parlamento, tra i diversi modi di vedere. Tali situazioni e tempi impongono una non frettolosa riflessione e possono determinare un confronto sensibile e approfondito, qualunque possa essere in definitiva la conclusione approvata dai più». Ritengo che questa sia la direzione lungo la quale muoverci, puntando ad una discussione franca, sciolta dalla tentazione di scivolare da entrambe le parti in una contesa politica che finirebbe con il danneggiare prima di tutto la nostra democrazia. Non dobbiamo lasciare prevalere lo stimolo di fare qualcosa a tutti i costi, a scapito della qualità di quello che bisogna realizzare e fare. A noi spetta la responsabilità di interpretare fino in fondo il ruolo di legislatori, scongiurando il rischio che il dibattito che si sta svolgendo sia fine a se stesso e la legge sul fine vita diventi un altro degli *spot* cui ci ha abitato il Governo Berlusconi, un'ulteriore pubblicità da trasmettere al Paese, magari in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali. Onorevoli colleghi, la vita e la morte non possono essere politicizzati, né su valori come il rispetto per la persona umana e la libertà di coscienza si può pensare di decidere a maggioranza. È scritto nella Carta costituzionale al troppo spesso citato, ma ancora poco studiato e conosciuto articolo 32. Certamente non viene colto da parte del legislatore il riferimento che si cita in questo articolo: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Il riferimento, anche in questo caso, su un argomento così delicato all'opera dei Padri costituente appare quanto mai mirabile e chiarissimo. A noi legislatori del XXI secolo spetta tradurre in atto normativo quell'indirizzo con l'obiettivo di formulare una legge seria, ragionevole e - mi permetto di aggiungere - ragionata e responsabile. Non possiamo confondere la nostra azione, il compito delicato ma affascinante che ci spetta con la fede o con il riferimento al pensiero laico. Lo dico da cattolico praticante. Oggi, guardando a quando sta accadendo nella discussione sul fine vita, ma anche in relazione ad altre questioni di interesse nazionale, mi sembra quasi che molti più che a servirli tendono a servirsi della Chiesa e dello Stato, confondendo i piani e le sfere di azione e di interesse, con riferimento alla crisi di valori e delle culture tradizionali e storiche. Riflettendo sulla contrapposizione, a mio avviso stucchevole e dannosa, che si sta alimentando da mesi sul testamento biologico, tra laici e cattolici, mi è tornata alla mente la straordinaria lezione di Sturzo. Sono passati novant'anni dalla pubblicazione, ma l'appello che egli rivolse agli "uomini liberi e forti" risuona come un richiamo altissimo. Non lasciamolo cadere come voce che grida nel deserto; noi uomini del nuovo millennio dovremmo tornare a sentirci liberi e forti cercando di mettere a frutto l'eredità del padre del popolarismo nel rispetto della sensibilità anche di culture diverse. Per Sturzo i cattolici dovevano impegnarsi in politica, ma tra politica e Chiesa doveva esserci assoluta autonomia. [**Presidenza può essere ispirata da princìpi cristiani, ma non si può tornare allo schematismo del passato. Questa è una straordinaria lezione di laicità nei tempi moderni. La religione può suggerire, ma non imporre. La religione - mi rivolgo ai cattolici democratici e a tutti coloro che quasi tirano per la tonaca la Chiesa e i vescovi - non può essere ridotta a strumento di Governo o di parte. vale per la religione cattolica e ovviamente per tutte le altre confessioni religiose. Il legislatore, pur non professando, in piena legittimità di scelta, ci mancherebbe altro, alcuna fede, ha il dovere di far rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini, così come evade dal suo ambito se, pur ispirato dalla propria confessione religiosa, non rispetta chi non mette la religione al centro delle proprie scelte. il motivo per cui ritengo poggi su basi erronee la discrasia troppo spesso alimentata strumentalmente tra laici e cattolici. I laici non sono un blocco rigido, non costituiscono un'anticonfessione opposta ai cattolici. La laicità non necessariamente prescinde dalla fede. È il motivo per cui ritengo che, posta in questi termini, la discussione del fine vita sia destinata a rimanere ancora monca, come nella proposta della maggioranza, allontanando inesorabilmente la possibilità di individuare una soluzione. Fede e laicità possono ritrovarsi sul terreno comune della ricerca, del dubbio, base portante di entrambi e, soprattutto, nella necessità di tutelare le aspirazioni di ogni singolo individuo. È l'individuo la base della socialità e di fatto esso viene prima della società, il che ci porta all'articolo 32 della Costituzione e alla necessità che esso, nella legge sul fine vita, non venga intaccato, come invece mi sembra accada con il disegno di legge del Governo. Non una legge che autorizzi a staccare la spina, dunque, ma una norma che garantisca a ciascuno la facoltà di scelta secondo coscienza. È proprio la coscienza l'unico riferimento. inutile imporre un regime militare e pretendere che su tali temi si possa obbedire ad ordini di scuderia. Bisogna garantire il diritto di ciascuno di decidere secondo la propria autonomia di scelta, come giustamente ha fatto notare più volte il segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini. Nella legge da formulare non può non essere accettato il principio per cui è l'individuo, nel suo essere persona, a decidere sui trattamenti attraverso la dichiarazione anticipata di trattamento. Ha ragione la presidente Finocchiaro quando, riferendosi all'emendamento del comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge, che ammette l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutrizione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, sottolinea: «L'idea che la legge obblighi il cittadino a subire determinati trattamenti - perché la nutrizione forzata attraverso sondini o tubi gastrici è un trattamento o l'idea che una persona possa essere obbligata dalla legge a subire trattamenti che non desidera, è un'idea che non ha uguali in nessun Paese civile». Con lei, anche noi ci auguriamo che agli italiani non venga riservato un tale trattamento. Ne va del rispetto dell'individuo, della civiltà di un popolo, della maturità della democrazia nel nostro Paese. Etica e princìpi, che sono il presupposto del rispetto della persona umana, l'uomo nella sua essenza, senza strumentalizzazioni e forzature politiche di parte, tra laici e cattolici, segno di una cultura e di una civiltà che ci fa essere una democrazia matura.

Dobbiamo avere il senso della responsabilità, anche rispetto ai tempi nuovi che si annunciano e anche rispetto a un mondo incerto, dove i valori e la decadenza civile rischiano di mettere in pericolo e in discussione il futuro della democrazia del nostro Paese.

Grazie il 19 marzo di sette anni fa, a pochi passi dalla sua casa di Bologna, sotto i colpi di una violenza politica che molti credevano ormai consegnata alle pagine più dolorose della storia del nostro Paese, cadeva barbaramente assassinato il professor Marco Biagi. Nella sua follia criminale, guidata da un cieco delirio ideologico, il terrorismo brigatista attribuiva a questo mite studioso, pioniere della comparazione giuridica in materia di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, una insanabile colpa. Quella di aver collaborato, tra il 1995 e il 2002, alle attività di tre Governi, di differente orientamento politico, mettendo a disposizione del Paese le sue eccezionali competenze e e contribuendo a realizzare quelle riforme del mercato del lavoro che la sua attività scientifica, instancabilmente divulgata anche al di fuori del mondo accademico, mostrava ormai come una esigenza indifferibile del nostro sistema produttivo. Questo tenace spirito di innovazione aveva trovato espressione nel Libro bianco sul mercato del lavoro significativamente intitolato «Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità», pubblicato, nell'ottobre del 2001, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'idea portante del Libro bianco era costituita appunto dall'idea, formulata in particolare da Marco Biagi, di procedere verso l'obiettivo della società attiva: un modello sociale e produttivo, cioè, radicalmente innovativo rispetto a quello sperimentato dal nostro Paese negli ultimi decenni. L'obiettivo, assai ambizioso, era quello di costruire un sistema in cui le ragioni della crescita economica e le esigenze della produzione potessero finalmente convivere con la qualità della vita personale e familiare dei lavoratori e, di conseguenza, con la crescita demografica ed il pieno sviluppo della persona umana. L'urgenza che si manifestava era quella di dare un'attuazione piena, adeguata all'evoluzione dei rapporti economici e sociali, alla disposizione dell'articolo 35, primo comma, della Costituzione, secondo la quale «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Per far questo occorreva però superare un meccanismo di tutela ingessato sulla difesa dei rapporti di lavoro esistenti, che lasciava senza alcuna protezione le tantissime posizioni di lavoro atipiche o precarie che proprio in quegli anni si erano diffuse fino a diventare una parte importante della realtà produttiva del nostro Paese. Di fronte alle critiche e alle accuse di chi vedeva nel progetto soltanto l'obiettivo di limitare i diritti e le tutele esistenti, il professor Biagi ribadiva (come fece anche poche settimane prima della sua morte, nel corso di un incontro con la Conferenza episcopale italiana) la necessità di considerare la sua proposta in tutti i suoi aspetti. Ad un aumento della flessibilità dei rapporti di lavoro si affiancava inscindibilmente, infatti, un significativo rafforzamento degli ammortizzatori sociali, degli incentivi per l'occupazione, degli interventi dei servizi pubblici e privati per l'impiego e soprattutto - ripeteva il professore - tutta la riforma si poneva in continuità con gli interventi avviati nella precedente legislatura dal Governo di centrosinistra. Un percorso riformatore, quindi, libero da qualsiasi matrice ideologica o di interesse, tratteggiato nelle sue priorità da quello che costituiva, in coerenza con la sua formazione di comparatista, il parametro fisso dell'analisi di Marco Biagi, cioè il suo guardare costantemente all'Europa, consapevole della necessità imprescindibile, per il sistema italiano, di restare al passo degli altri partner europei. Al di là dei contenuti e delle proposte, la vita e l'azione di Marco Biagi possono offrire ancora al mondo della politica e delle istituzioni due preziosi contributi: in primo luogo, la sua fiducia nel dialogo come strumento privilegiato per la modernizzazione del Paese, che non può realizzarsi compiutamente se non attraverso il convincimento e la consapevolezza di tutti i principali attori del cambiamento. Il considerare che la voce di quest'uomo del dialogo sia stata spenta dall'antitesi del dialogo stesso, cioè dall'intolleranza ideologica che si fa violenza e terrore, non fa che aggiungere a questa qualità una vena di testimonianza profetica. È compito di tutti noi, oggi, raccogliere questa testimonianza. Traspare poi, in tutti i suoi contributi, una solida fiducia nel ruolo insostituibile delle istituzioni democratiche, come luogo di sintesi dell'interesse generale, che si alimenta dal confronto con gli interessi particolari rappresentati dalle parti sociali, ma non è mai asservito ad essi. Anche se ha conseguito una prima, organica realizzazione con la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, significativamente ribattezzata da tutti i commentatori con il nome di «legge Biagi», quel prezioso bagaglio di idee e di proposte attende ancora una più compiuta attuazione. Penso, in particolare, alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono ancora, nel nostro Paese, un diffuso ricorso al lavoro a tempo parziale, che nell'analisi del professore bolognese costituirebbe una delle più efficaci soluzioni per migliorare i tassi di occupazione femminile e giovanile ancora tra i più bassi d'Europa - e per compiere un altro significativo passo in avanti verso l'obiettivo della società attiva, dando attuazione, nello stesso tempo, all'articolo 37 della Costituzione, che impone che le condizioni di lavoro consentano alla donna lavoratrice «l'adempimento della sua essenziale funzione familiare». Il coraggioso riformismo del professor Biagi, sostenuto dalla mirabile lucidità della sua analisi, avrebbe senza dubbio costituito oggi una preziosa risorsa per la politica e per le istituzioni, nel difficile contesto economico e sociale del nostro tempo, marcato da crescenti effetti sull'economia reale di una crisi finanziaria di proporzioni globali. Oggi di lui ci resta il ricordo: è per noi dovere di continuare ad attingere al suo prezioso patrimonio di idee con spirito di dialogo, per non rendere vano il sacrificio di un uomo che al progresso dei lavoratori e della società civile ha dedicato la propria vita.

chiedo scusa a lei e a tutti i colleghi se non potrò ascoltare le considerazioni che alcuni di loro vorranno svolgere in ricordo di Marco Biagi. Purtroppo devo lasciare l'Aula per raggiungere Bologna per uno degli appuntamenti che ogni anno da sette anni a questa parte si svolgono per ricordare Marco Biagi. Tra questi segnalo quello che che usualmente si svolge a Modena, presso la sua università, alla quale era molto legato, alla presenza autorevolissima, quest'anno, del Presidente della Repubblica. Modena opera la fondazione a lui dedicata, che Marina Biagi volle quella sera stessa e che ha nel professor Tiraboschi, che ne ha preso la cattedra, il suo animatore. Ricordo quando, pochi giorni prima di quella maledetta sera, egli mi disse che, qualunque cosa gli fosse successa, aveva organizzato tutto affinché potessi ancora essere assistito nel completare quel percorso, perché il professor Tiraboschi era in grado di sostituirlo in tutto e per tutto. In effetti Marco Biagi era un uomo generoso, non era un docente geloso del suo sapere. Aveva una grande capacità di coinvolgimento nei confronti dei suoi allievi che anche oggi sono uniti da un rapporto solidale nella stessa fondazione e nel centro studi da lui fondato. hanno proseguito il suo lavoro, in modo particolare per quanto riguarda la rete dei rapporti internazionali che egli aveva avviato, una rete che ne faceva, forse caso unico, un ottimo comparatista in una materia, quella del diritto del lavoro, che usualmente rimane gelosamente chiusa nella dimensione nazionale, come se dovesse essere solo espressione della specifica storia di un Paese, della storia delle sue relazioni industriali e non invece parte di quei confronti competitivi che sempre più includono

soprattutto il suo orientamento alla società attiva. Non era certamente un docente di diritto del lavoro né ideologizzato né autoreferenziale, non si accontentava della pulizia formale della norma, odiava anzi il formalismo giuridico. Potremmo dire che era soprattutto un uomo ansioso di risultati, di risultati, che egli cercava soprattutto nell'inesorabile verifica che dà l'andamento del tasso di occupazione, misura non esclusiva ma certo fondamentale per comprendere il grado di attività di una società, la sua capacità di essere inclusiva e allo stesso tempo competitiva, perché appunto capace, includendo, di apprezzare il proprio capitale umano. Lei, Presidente, ha altresì segnalato come la legge che porta il suo nome costituisca un giacimento in parte ancora inespresso, vi siano cioè in essa molte intuizioni che meritano maggiore impegno per darvi attuazione. Ha citato opportunamente la modulazione dell'orario di lavoro, che consente una maggiore conciliazione fra tempi di lavoro e di non lavoro. Aggiungo la piena attuazione di quei contratti di apprendistato che Marco Biagi volle per salvare una generazione di giovani di cui egli individuava la patologia dell'uscita tardiva da percorsi formativi spesso troppo deboli per essere apprezzati dal mercato del lavoro.

si possano dire superate, sulla base di prese di posizione autorevoli che vi sono state, quelle lacerazioni che ne hanno accompagnato il lavoro. Ma questo è spesso il destino dei riformisti:

Signor Presidente, colleghi senatori, sette anni fa la furia omicida del terrorismo brigatista colpiva il giuslavorista Marco Biagi, sotto la sua abitazione, in via Valdonica, a Bologna. L'odio cieco ma mirato della violenza terroristica ha tolto al nostro Paese un professionista apprezzato, un vero intellettuale, un esponente della migliore cultura riformista dell'Italia. Oggi, il professor Biagi è noto soprattutto per la sua legge sul mercato del lavoro; ma è doveroso ricordare che la sua grande competenza lo rese "immune" da qualsiasi vicinanza o affiliazione partitica: lavorò indistintamente per Governi di diverso colore politico, fu consulente del CNEL e la sua attività fu stimata ed apprezzata anche in sede europea. Il suo obiettivo più ambizioso, infatti, era una riforma complessiva del sistema sociale ed economico del nostro Paese, che potesse partire dal nodo centrale del mercato del lavoro. Biagi capì c'era bisogno di una scossa: in particolare, tra i tanti aspetti critici, trovò nell'eccessivo costo del lavoro il vero motivo dell'enorme disoccupazione di quel periodo nel nostro Paese. Un'evidente difficoltà per i giovani nel trovare un posto di lavoro, che si trasformava presto in rassegnazione alla disoccupazione o nella ricerca di forme inadeguate, non tutelate né regolarizzate e quindi illegali di impiego. C'era bisogno di una riforma che prendesse di petto i problemi. «In Italia» - notava giustamente Biagi - «abbiamo il peggior mercato del lavoro d'Europa» e «non vi sono davvero alternative. Ignorare le richieste di modernizzazione (...) sarebbe in fondo una scelta egoistica, propria di chi pensa a se stesso e non immagina un futuro migliore per i propri figli». Animato da questi propositi, diede vita a quella riforma che oggi prende proprio il suo nome: una legge che è stata oggetto di molti apprezzamenti, compresi quelli del nostro partito, ma anche di aspre critiche. Sulla flessibilità del lavoro e sugli effetti che la «legge Biagi» ha portato nella nostra società, molto si è detto. C'è chi la considera l'anticamera del precariato, chi invece l'unica concreta possibilità per chi non ha un impiego. Una cosa è certa: il professor Biagi ha saputo interpretare un'esigenza di fondo della nostra società, quella della flessibilità del lavoro, unico antidoto alla disoccupazione, unica soluzione per rimanere agganciati al treno dell'Europa e poter competere con i nuovi mercati mondiali e la loro estrema competitività. Grazie al professor Biagi, la preparazione e le capacità dei più giovani potevano finalmente esprimersi ed essere valutate. Con loro, anche gli stessi datori di lavoro venivano finalmente responsabilizzati, e portati a proporre alle nuove leve regolari contratti di inserimento, che poi sarebbero potuti sfociare in assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Una possibilità reale, quindi, per tante persone finora messe alla porta dalle regole del lavoro, ma anche per le aziende, per le molte piccole e medie imprese che si sentirono "capite" da questa legge e che grazie ad essa sono riuscite ad innovare, ad investire, a dare fiducia alle nuove generazioni senza cadere nella tentazione di spostarsi all'estero. Inutile ricordare che le tesi di Marco Biagi, così innovative e rivoluzionarie, lo resero un personaggio scomodo politicamente e, purtroppo, un obiettivo sensibile per il terrorismo. La sua unica colpa, infatti, era quella di cercare soluzioni diverse da quelle care a una certa matrice estremista. Venne assassinato dalla mano vigliacca e impaurita di chi elimina fisicamente perché non sa contrapporre idee. Il suo omicidio deve farci anche riflettere sulla drammatica attualità del terrorismo interno, la cui fiamma antagonista non si è spenta ed è alimentata da quella cultura dell'odio e dell'emarginazione che ancora oggi è presente nel nostro Paese. Oggi, per fortuna, di Marco Biagi ci resta molto: una legge di stampo liberale, appunto, ma anche un modello di riformismo coraggioso da seguire, da imitare e da attuare integralmente soprattutto in questo periodo di crisi economica e finanziaria. Ci restano le sue parole, mai banali, quelle che ricordavano a tutti, anche ai più sordi, di non aver paura delle riforme, di cercare in tutti i modi di migliorare la nostra legislazione per una "società più giusta". Signor Presidente, colleghi senatori, Marco Biagi è una persona morta sul lavoro e uccisa per il suo lavoro. Oggi, a sette anni di distanza dalla sua morte, ricordiamo una persona che venne assassinata perché ebbe il coraggio di proporre cambiamenti. Perché forse il suo vero grande obiettivo era quello di dare ai giovani, a quei giovani dai quali ogni giorno si dirigeva in bicicletta per fare lezione, non solo tanti utili insegnamenti, ma anche una concreta speranza per il futuro. Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento vorrei davvero esprimere il mio apprezzamento per il suo intervento, per la cura che ha avuto nel ricostruire la vicenda e per la sensibilità istituzionale che l'ha caratterizzato. Credo che esso sia la cornice migliore per le nostre riflessioni. II 19 marzo di sette anni fa le Nuove Brigate Rosse uccidevano a Bologna il professor Marco Biagi. Erano le stesse Brigate Rosse che avevano colpito mortalmente Ezio Tarantelli il 27 marzo del 1985 e poi Roberto Ruffilli il 16 aprile del 1988 e Massimo D'Antona il 20 maggio del La morte di un uomo, di qualsiasi uomo in qualunque luogo e per qualunque ragione, è una tragedia irreparabile. Niente può renderle ragione, come niente può colmare il vortice di vuoto che una morte crea nell'universo attraversato da colui che è stato una vita. In più, negli omicidi terroristici c'è sempre una componente simbolica che si aggiunge alla terribile volontà distruttiva delle vite umane. E così è stato anche per Marco Biagi. Il professor Biagi forniva il suo importante contributo intellettuale e professionale alla gestione del processo di cambiamento dell'economia globale e delle regole del mercato del lavoro che da quella trasformazione discendono. La sua era dunque una delicata funzione di cerniera tra lo Stato e la società nelle sue articolazioni. Una funzione rivolta a costruire un nuovo quadro di riferimento normativo e legislativo. Il suo era un lavoro svolto da consulente dei Ministeri dei diversi Governi che si sono succeduti e rivolto principalmente alle forze sociali, ai loro rapporti, al merito che le stesse affrontano quotidianamente. Il lavoro del professor Biagi era dunque destinato a costruire un tessuto di relazioni in grado di ridurre il potenziale conflitto che i cambiamenti profondi della società e dell'economia possono stimolare.

In quel momento davvero era delicatissimo affrontare quelle tematiche. La cosa tragica era che noi tutti pensavamo che quella spirale si fosse conclusa, quando invece la mano omicida delle Brigate Rosse colpì il professor D'Antona e il professor Biagi. professor Biagi. Il mio ricordo personale è di grande gratitudine per il professor D'Antona, che ho avuto la fortuna di conoscere, e certamente nella stessa linea si inserisce il mio sentimento nei confronti del professor Marco Biagi. Ezio Tarantelli aveva realizzato sulla regolazione della redistribuzione dei redditi, e per il quale Roberto Ruffilli si era occupato per i temi della riforma delle istituzioni, con grande anticipo sui tempi. È questo filo di responsabilità forte che la follia dei terroristi ha voluto recidere. Al professor Biagi si deve il Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia e rivolto al contrasto dell'economia sommersa, per più occupazione e meno precarizzazione, contro il lavoro irregolare e clandestino che contribuisce a creare condizioni di esclusione sociale. Quanto torto si è fatto al professor Biagi nella ricostruzione faziosa delle sue iniziative in questa materia, davvero grandi torti! In quel testo, ad un certo punto, si legge: «Le esperienze dei paesi europei che hanno con più successo riformato il mercato del lavoro, mostrano quanto sia importante disporre anche in Italia di un nuovo assetto della regolazione e del sistema di incentivi e ammortizzatori, che concorra a realizzare un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza. Tale sistema deve avere come obiettivo ultimo quello di accrescere l'occupazione e di diminuire le forme di precarizzazione». Questo era l'obiettivo per il quale Marco Biagi ha lottato. E la sua barbara uccisione ci riconsegna ogni anno, intatta, la riflessione sulla sua opera e sulla sua figura. Rileggere oggi il Libro bianco ci aiuta a comprendere la portata del lavoro del professore bolognese e la qualità della sua proposta. Le sue doti di studioso sicuramente attestate dai numerosi e importanti scritti che, con rigore di metodo e sempre con raffinato tecnicismo, hanno se non preceduto, e, comunque, hanno consolidato i momenti più significativi dell'evoluzione del diritto del lavoro degli ultimi venti anni. Le sue scelte, come è necessario per un intellettuale, sono sempre state precise scelte di campo: egli ha sempre proposto interpretazioni della legge che consentivano una più intensa ed effettiva tutela di chi lavora. E che queste interpretazioni siano state proposte con rigorosa coerenza di metodo, e quindi con equilibrata consapevolezza, non significa affatto che comportassero ipotesi di mediazione. Anzi, proprio quelle interpretazioni hanno finito per alimentare il dibattito necessario anche al progresso della scienza giuslavoristica. In quel lavoro Marco Biagi vedeva quasi una nuova utopia, un nuovo compito per il sindacato, la capacità di ricollegare la difesa del valore di mercato del lavoro, la quantità del lavoro, alla sua qualità, a quello che significa per la persona in carne ed ossa che lavora: riconnettere il valore di mercato del lavoro alla soddisfazione, alla motivazione, alla realizzazione di sé che una persona nel lavoro può trovare. Un'utopia, quella di Biagi, che mi ricorda l'operaio specializzato Faussone nel libro «La chiave a stella» di Primo Levi: quando ad un certo punto gli chiedono che cos'è la felicità, risponde che non sa che cos'è la felicità, ma che «fare un lavoro che ti piace, farlo bene è la cosa che si avvicina dì più». Ecco, Marco Biagi era una persona che faceva un lavoro che gli piaceva e lo rendeva felice. Da questo punto di vista, uccidere una persona felice è un crimine ancor più grave e più pesante. Ricordare in questa solenne aula il professor Biagi e il suo sacrificio, significa guardare anche alla necessità assoluta di escludere la logica della violenza dalle dinamiche di ogni lotta e dal quotidiano. C'è la necessità assoluta di ricordare, che deve essere integrata da quella di indagare, scoprire, conoscere. Il terrorismo, rosso e nero, a sfondo politico o religioso, è una malattia che va debellata, anche nel nostro Paese. Deve essere trovato un vaccino, che parta dalle scuole, dai posti di lavoro, dai diritti e dai doveri, dalle libertà. Questo vaccino, per essere iniettato, ha bisogno di un supporto culturale, ha bisogno di una conoscenza più diffusa. Si deve sapere per non ripetere, per non permettere che cali la nebbia sulle vittime e sui meccanismi che, nel tempo, hanno portato persone a credere nel potere della violenza e a vedere nello Stato e nelle istituzioni un bersaglio anziché una garanzia. Gli anni di piombo che hanno segnato la storia del nostro Paese, così come l'attentato al professor Biagi, fanno parte di un passato che non deve più tornare, ma che non si deve nascondere o recludere nell'oblio storiografico. L'ideologia di morte va estirpata. Va abbattuta definitivamente e, proprio per questo, la memoria è importante per fare da ponte tra passato, presente e futuro, per cambiarli, per permettere che siano migliori. Questo barbaro omicidio di matrice terrorista compiuto sette anni fa, e gli altri che tragicamente lo hanno preceduto, ci mandano a dire che il nostro Paese dovrebbe essere unito sui valori e i princìpi di fondo. Deve esserlo oggi come lo è stato vent'anni fa quando la violenza terroristica toccò il suo apice. Credo che questo, e non altri, è il vero banco di prova della nuova classe dirigente. Se ripartiamo da qui, da questa volontà, non solo saremo più forti nella lotta al terrorismo ma onoreremo al meglio la memoria di chi, come Marco Biagi, è caduto per le sue idee e per la loro difesa. *(Applausi)*. Signor Presidente, fu un omicidio terribile quello che ci portò via Marco Biagi il 19 marzo del 2002. Terribile perché l'agguato terroristico di cui rimase vittima, ad appena 51 anni, colpì le coscienze di tutti gli italiani sinceramente democratici. Fu terribile perché ci riportò di colpo indietro ad anni funesti, che pensavamo di esserci lasciati alle spalle, ma di cui qualche tempo prima avevamo avuto un primo rigurgito con il vile assassinio di un altro insigne giuslavorista, Massimo D'Antona, meno di tre anni prima, nel giugno del 1999. Terribile perché pensavamo che quella sigla, quella delle Brigate Rosse, fosse ormai passata alla storia e che nel 2002 fosse ormai fuori dalla storia; invece ce la ritrovammo nella cronaca, tragicamente. Ma quel feroce assassinio fu terribile anche perché ebbe strascichi polemici e la sua famiglia, ancora oggi, non partecipa a commemorazioni ufficiali. Biagi aveva chiesto con insistenza, proprio nelle settimane precedenti il suo assassinio, che gli fosse di nuovo assegnata una scorta. Non sappiamo se questo avrebbe convinto i suoi assassini a desistere dall'agguato. Sappiamo però che è morto solo, sotto casa sua a Bologna, e che un po' di buon senso da parte di chi allora avrebbe dovuto decidere sull'assegnazione della sua scorta avrebbe dovuto indurre lo Stato ad una maggiore protezione dei suoi migliori servitori, uno dei più esposti. E che fosse uno dei più esposti lo si sapeva, almeno dal maggio del 1999. Oggi è il tempo della memoria. Ricordiamo un giuslavorista pignolo, coscienzioso, preciso nelle sue considerazioni, moderno, nell'accezione migliore del termine, che aveva studiato, grazie anche agli incarichi che gli erano stati assegnati, il mercato del lavoro a livello globale. Nel 1997 era stato rappresentante del Governo italiano nel comitato dell'Unione europea per l'occupazione e il mercato del lavoro. ancora, aveva ricoperto altri incarichi, a livello italiano ed europeo, senza mai lasciare la cattedra di diritto del lavoro, che esercitò a Pisa, all'Università della Calabria, a Ferrara, a Modena, a Reggio Emilia. Dopo l'esperienza all'Unione europea divenne consigliere dei Ministri del lavoro dei Governi Prodi, D'Alema e Amato. Quando nel 2001 Berlusconi vinse le elezioni, Biagi fu confermato consigliere dall'allora ministro dell'interno Maroni, segno della terzietà e dell'imparzialità delle sue indagini. Insomma, Biagi era una di quelle persone senza le quali fare una riforma diventa più difficile, uno dei maggiori esperti di lavoro in Italia e in Europa. Oggi è il giorno della memoria, dicevo, non della polemica. Voglio solo - ma lo dico con pacatezza - aggiungere che probabilmente Biagi non si sarebbe nemmeno intestato la legge a cui hanno dato il suo nome, la n. 30 del 2003. Andando a rileggere i suoi scritti, i suoi studi, non tutto quello che è stato riportato nella legge n. 30 corrisponde alla volontà del giuslavorista bolognese. Biagi conosceva benissimo il mercato del lavoro e la sua globalizzazione, la sua internazionalizzazione. Un sistema ingessato, come quello italiano fino a metà degli anni Novanta, aveva bisogno di una riforma incisiva. Ed è quello che aveva fatto il centrosinistra con la legge n. 196 del 1997, che aveva introdotto in Italia le prime norme sulla flessibilità. Il Governo Berlusconi, che aveva vinto le elezioni nel 2001, aveva subito iniziato l'*iter* che avrebbe poi portato alle legge n. ma il Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia di Biagi, pubblicato proprio nel 2001, era rivolto, cito, «al contrasto dell'economia sommersa», e contro il lavoro «irregolare e clandestino che contribuisce a creare condizioni di esclusione sociale». Insomma, Biagi voleva - lo cito ancora - «più occupazione e meno precarizzazione». Quello che il centrodestra con la legge n. 30 non ha fatto è stato proprio creare una serie di contrappesi e di garanzie sociali che nei libri di Marco Biagi c'erano ed erano anzi indispensabili per la buona riuscita della riforma. Un precario che perde il posto di lavoro ha bisogno di un paracadute che il Governo Berlusconi, in nome di una ideologia liberale di stampo thatcheriano e più in generale anglosassone, già fallita miseramente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, ha voluto deliberatamente escludere. Biagi aveva studiato il diritto del lavoro dei principali Paesi europei e arrivava alla conclusione di quanto fosse «importante disporre anche in Italia di un nuovo assetto della regolazione e del sistema di incentivi e ammortizzatori» per concorrere «a realizzare un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza». «Tale sistema» - scriveva ancora Biagi - «deve avere come obiettivo ultimo quello di accrescere l'occupazione e di diminuire le forme di precarizzazione». Se qualche risultato nella crescita dell'occupazione in questi anni si è avuto, la sicurezza del lavoro è ancora oggi un'opera incompiuta. Fino a ieri, dicevo, perché oggi la situazione sta drammaticamente peggiorando a causa della crisi economica. Altro che sicurezza, altro che tutele, altro che flessibilità. I precari oggi sono i più colpiti dalla crisi e la percentuale di occupati sta inesorabilmente diminuendo. Io credo che questo sia il momento di andare a rileggere le pagine scritte da Biagi e, se proprio si vuole fare fino in fondo onore alla sua memoria, si porti a compimento la sua opera integralmente, non solo in parte. Stiamo chiedendo con forza una riforma degli ammortizzatori sociali. In questo momento, per superare la crisi, bisogna aiutare i più deboli, quelli che il lavoro lo hanno perso o lo perderanno nei prossimi mesi. Di questo equilibrio tra flessibilità e sicurezza Biagi parlava già nel 2001. Basta ascoltarlo. *(Applausi).*

siamo oggi in quest'Aula a ricordare il settimo anniversario del vile e criminale assassinio di Marco Biagi, avvenuto in silenzio, una sera come tante in cui tornava a casa dopo infaticabili giornate di studio e lavoro. Ma oggi siamo qui soprattutto a ricordare la sua vita, la vita e il pensiero di una figura di spicco del mondo politico e giuslavorista, di colui che diede la propria vita per garantirne una diversa alle nostre lavoratrici e ai nostri lavoratori, ai nostri figli, e per offrire loro un futuro e quel senso vero di autostima che dà il lavorare. Socialista e cattolico, Marco Biagi si era posto il problema di come modernizzare il mercato del lavoro ed era culturalmente ben preparato, dopo numerose esperienze come professore universitario e come consulente di diversi Ministri del lavoro di entrambi gli schieramenti. Da buon conoscitore del diritto del lavoro nazionale e internazionale invocava la comparazione con gli altri ordinamenti ed è grazie anche alla sua opera se oggi nel nostro Paese abbiamo una normativa moderna e ben fatta, delle più avanzate a livello europeo. Lo si deve in gran parte alla «legge Biagi», che ha creato in questi anni molti posti di lavoro e ha regolato il lavoro precario, settore in cui non c'erano regole. Marco Biagi ci ha lasciato una grossa eredità: tutti quelli che si occupano delle questioni che lui ha così appassionatamente seguito, quelli che lo hanno conosciuto o lo hanno letto, o quelli che semplicemente si sono interessati alle politiche del lavoro non possono prescindere dal suo pensiero. Non possono non ricordare con quale forza d'animo e d'intelletto agiva e pensava per creare delle riforme per il bene del nostro Paese, per far sì che questo non soccombesse a causa della forte competitività con gli altri Paesi europei. Biagi era uno degli autori del Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, un documento di proposte concrete e serie, in cui tra l'altro si definiva che ciò che deve essere salvaguardato non è tanto il valore assoluto della retribuzione, bensì il suo reale potere di acquisto. In quel testo era condensata tutta la filosofia del cambiamento, teso a portare regole nuove del mercato per creare una società moderna e al passo coi tempi. E in questo Marco Biagi, anche se proveniente da una diversa area culturale, aveva condiviso la spinta sociale e riformatrice di cui la Lega Nord è protagonista. I colpi di pistola che hanno spezzato la breve vita di questo uomo dai modi gentili, sempre pronto al dialogo e alla mediazione, hanno voluto mandare un segnale terribile: non provate a cambiare, a far uscire il Paese dalla burocrazia e dall'immobilismo del sistema. E invece no. Bisogna avere il coraggio di fare le riforme, le riforme che ci chiede la nostra gente e che sono necessarie al nostro Paese. Anche in nome del sacrificio di Marco Biagi, cambiare è sempre più un dovere. Bisogna continuare con il processo riformista, non solo nel mondo del lavoro. E il dialogo è la migliore risposta che si possa dare a chi si oppone ai cambiamenti. Tutti dobbiamo andare avanti sulla strada di un confronto costruttivo, fuori dagli schemi ideologici e di contrapposizione tra i diversi schieramenti. Bisogna evitare strumentalizzazioni e cercare invece di fornire le risposte alla nostra gente, al mondo del lavoro e alle imprese che si trovano, soprattutto ora, ad affrontare un periodo di crisi molto, ma molto delicato. Le riforme vanno assolutamente affrontate senza pregiudizi e senza esasperare gli scontri o i toni del dibattito. Agli occhi dei terroristi, delle Nuove Brigate Rosse, la "colpa" di Marco Biagi era quella di essere un riformista che lavorava anche per il Governo Berlusconi e per il ministro Maroni; un uomo tenace ed ostinato nell'andare avanti con la coerenza delle proprie idee senza arrendersi. Non si può morire per questo. Il terribile omicidio di Marco Biagi ci dovrebbe far riflettere in tal senso e vi assicuro, cari colleghi, che una mattina, pur avendo scoperto di essere anch'io in quell'elenco, non ho avuto paura e sono andata avanti. Anche Marco Biagi non ha avuto paura ed è andato avanti a lavorare. Per me, che ho avuto la fortuna di conoscerlo al tavolo delle trattative, è un onore ricordare oggi in quest'Aula Marco Biagi. Certi Certi avvenimenti e certi insegnamenti vanno ricordati sempre e, anche dopo la morte, il pensiero di uomini come Biagi deve essere sempre vivo nella società.

Qualcuno ha ritenuto di contrapporre il pensiero dell'uno a quello dell'altro e, certo, tra l'uno e l'altro è facile ravvisare differenze anche marcate su singoli punti. Entrambi erano però animati da una convinzione, che, a ben vedere, è assai più rilevante di quelle differenze; una convinzione che non è di per sè né di destra, né di sinistra, ma è soltanto profondamente ragionevole: la convinzione, cioè, secondo cui il diritto del lavoro può essere difeso efficacemente soltanto se lo si aiuta a evolvere, ad adattarsi al mutare dei tempi, per poter conservare la propria essenziale funzione. L'uno e l'altro - Massimo D'Antona e Marco Biagi - in modi diversi hanno dedicato interamente la loro vita a questo mutamento

Sì, perché le Brigate rosse - le nuove come le vecchie - sono soprattutto una forza di conservazione. Nonostante i toni rivoluzionari del loro linguaggio, esse sono in realtà abbarbicate al vecchio ordinamento, lo difendono con le unghie e con i denti: i loro proclami, espliciti o impliciti che siano ("Lo statuto non si tocca", "Chi tocca l'articolo 18 muore"), sono la quintessenza del conservatorismo. Le Brigate rosse odiano chiunque lavori per la riforma del diritto del lavoro e per il suo adeguamento al nuovo contesto economico e sociale. Per questo i terroristi conservatori hanno puntato le loro armi contro Marco e Massimo e, prima di loro, contro Tarantelli, Tarantelli, Giugni, Ruffilli e tanti altri riformatori. La loro logica mafiosa - quella del "colpiscine uno per educarne cento" - era volta essenzialmente a paralizzare l'intelligenza riformatrice dell'intera comunità degli studiosi dei problemi del lavoro. La lezione di Marco Biagi, com'è stato sottolineato dal Presidente in apertura stamattina, e poi dal ministro Sacconi, è stata soprattutto una lezione comparatistica: le idee-forza che innervano il suo disegno *de iure condendo* nascono soprattutto dall'impegno a confrontarsi provinciali con tutte le esperienze offerte dal panorama internazionale, in particolare da quello nord-europeo. È da questo confronto che Marco ha tratto la convinzione dell'arretratezza, dell'iniquità, dell'inefficienza del nostro mercato del lavoro. Non me ne voglia il ministro Brunetta, che nei giorni scorsi ha invece ritenuto di qualificare questo nostro mercato del lavoro come "mirabile", "efficiente"; addirittura si è spinto a dire "equo". No, Marco era proprio convinto che questo mercato del lavoro fosse arretrato, iniquo e inefficiente; ed era convinto che ciò fosse conseguenza delle caratteristiche del nostro vecchio sistema di protezione e che per tale ragione questo sistema dovesse essere profondamente riformato. La legge che oggi porta il suo nome non esaurisce affatto il disegno complessivo che Marco aveva in mente negli ultimi tempi della sua esistenza. Quella legge, presentata da destra come la "grande liberalizzazione", quella che avrebbe dovuto "fare del nostro diritto del lavoro il più libero e liberale d'Europa", presentata da sinistra come "lo smantellamento del diritto del lavoro", non era in realtà né l'una cosa né l'altra: era soltanto un primo atto di razionalizzazione del mondo dei cosiddetti lavori atipici. Quando però Marco qualificava il nostro come "il peggiore mercato del lavoro d'Europa", e ne attribuiva la causa all'arretratezza del nostro sistema di protezione del lavoro, quella a cui pensava non era soltanto la razionalizzazione dell'esistente, bensì una vera e propria - uso le sue parole - transizione del nostro Paese dal vecchio equilibrio mediterraneo a un nuovo equilibrio di tipo nord-europeo. Una transizione di cui egli stesso aveva individuato i primi segni nella legislazione della seconda metà degli anni Novanta, in particolare nelle leggi del 1997, promosse dall'allora ministro del lavoro Tiziano Treu, e nella nota sentenza della Corte di giustizia che ci impose il superamento del monopolio statale nei servizi al mercato del lavoro. A proposito di questa transizione, vorrei che ascoltaste queste parole: con l'evoluzione verso il modello nord-europeo «il diritto al lavoro perde qualcosa rispetto ai densi riferimenti storici che lo connotano;» e questo qualcosa «è il forte orientamento all'avere, alla stabilità, all'uniformità. Avere il lavoro, ossia il posto, con le garanzie della inamovibilità, cosa che si può esprimere anche in termini di *property in job*... rimanda a un modello di impresa e di organizzazione del lavoro rigida, uniforme, durevole; un modello che tende al declino». Bene, queste non sono parole di Marco Biagi: sono parole di Massimo D'Antona; parole pronunciate nel suo ultimo intervento pubblico, 12 giorni prima che egli venisse ucciso. vedete, colleghi, come queste parole esprimono anche, con una straordinaria profondità e precisione, proprio la direzione nella quale si muoveva la riforma pensata da Marco Biagi e che andava al di là della sua stessa legge. Proseguo in quella citazione: «Il diritto al lavoro sembra spostare il suo baricentro sull'essere, ossia sulla persona. Quando si parla di impiegabilità della persona del lavoratore - il valore dell'*employability* sottolineato in tanti documenti comunitari quando si sottolinea l'irrinunciabilità di una tutela che assicuri a chi cerca, o cerca di conservare, il lavoro, uguali punti di partenza ma non uguali punti di arrivo, quando si indica nelle strategie di sostegno del lavoratore nel mercato il meglio che l'approccio microeconomico possa fare ... altro non si fa che prendere sul serio il diritto al lavoro come garanzia costituzionale della persona sociale, aggiornandola, però, come garanzia dell'essere e non dell'avere». Ancora una volta parole di Massimo D'Antona, che si combinano perfettamente per questo aspetto con l'idea di fondo di Marco Biagi. Questo dunque era, pur con le differenze innegabili sugli itinerari da percorrere ai quali ciascuno dei due pensava, il loro disegno di transizione. Oggi tocca a noi proseguire su quella strada. Per farlo dobbiamo innanzitutto spogliarci, gli uni e gli altri, di quel tanto di faziosità che sovente avvelena i nostri discorsi quando si parla di problemi del lavoro. Ma dobbiamo anche avere ben chiaro il senso profondo del declino irrimediabile del vecchio modello di protezione cui entrambi, Massimo e Marco, hanno cercato di dare uno sbocco positivo, al prezzo della loro vita. «Prendere sul serio il diritto al lavoro, come garanzia dell'essere del lavoratore» - di tutti i lavoratori, come lei stesso Presidente ha sottolineato all'inizio - «e non come diritto di proprietà su di un determinato pezzetto del tessuto produttivo» è l'essenza dell'esortazione che entrambi ci rivolgono. Forse abbiamo ancora qualche blocco mentale da superare, prima di riuscire a entrare davvero in questo ordine di idee, se ancora oggi,

dei vecchi assetti del sistema di protezione, del regime di *apartheid* che oggi in Italia segrega tra loro protetti e non protetti. A sette anni dalla morte di Marco Biagi e a dieci anni dalla morte di Massimo D'Antona, è tempo che, rispetto ai blocchi mentali del passato recente, voltiamo tutti pagina.

il mio primo incontro con Marco - lo ricordo benissimo - fu nella primavera del 1993. Gino Giugni ci aveva chiamati entrambi a far parte di una commissione ministeriale per la riforma dell'orario di lavoro. Ne nacque subito, istintiva, aperta, amicizia che ben presto divenne profondo patto professionale. Insieme lavorammo alla costruzione di nuove figure contrattuali, a cominciare da quel contratto "a chiamata" che sarebbe divenuto uno degli assi più densi della legge che, compiutamente e giustamente, al suo nome si intitola. E lungamente lavorammo intorno a quel modello partecipativo che Marco riteneva assolutamente essenziale nel momento in cui strategicamente il *foc**us* del modello di contrattazione si concentrava sul livello aziendale, perché, accanto e a fronte di questo accostamento, soltanto l'intensificazione della qualità cooperativa del lavoro ai fini del bene comune dell'impresa poteva dare compiuto orizzonte di senso a quel percorso.

cerca di stare più attento». Marco mi rispose con una forza e una nitidezza straordinarie, dicendomi: «Io non cambierò nemmeno il più piccolo dei miei gesti. Io non mi guarderò mai intorno quando poggerò la mia bicicletta al muro della stazione di Bologna perché,

alla setta oscena degli assassini, degli ultimi vili demoni del più oscuro Novecento. Ad un tratto, come rasserenandosi, mi disse: «Maurizio, è tempo che i professori, i manager e gli intellettuali si rimbocchino le maniche, si sporchino le mani, indipendente dagli schieramenti, dalle appartenenze, dalle sette, dai clan. Mettiamoci all'opera, mettiamoci tutti insieme a lavorare per costruire un mercato del lavoro più aperto, più giusto e più equo, un posto dove finalmente i giovani, le donne, gli anziani trovino un compiuto destino di dignità nel lavoro; dove un sistema competitivo non può essere tale se non è un sistema giusto. Un sistema non può essere giusto se non offre più ampiamente e riccamente opportunità, se non premia e non valorizza il merito, se non incorpora l'audacia delle prospettive e dei progetti». progetti». Vedendo poi i risultati degli anni a venire, osservando quel Paese il cui PIL non sapeva aumentare, ma che sapeva far crescere i suoi tassi di occupazione, ho capito quanta ragione avesse avuto Marco E quanto ancora, Presidente, come lei ha lucidamente osservato, avremmo bisogno di lui, della sua tensione, della sua visione progettuale, della sua capacità di innovare rinvenendo sempre i percorsi meno consueti e le traiettorie più intentate, da un lato, e, dall'altro, di quel suo pragmatismo anglosassone, curioso e saggio. Presidente, io, che a quel discorso devo il fatto di essere qui e che prego tutti i giorni di non essere indegno di quel maestro mite e coraggioso, non posso non considerare davvero quanto bisogno in questi tempi lacerati avremmo tutti anche del suo stile sobrio, quasi scabro, composto, quasi riservato, eppure capace di esprimere una repubblicana solennità solennità e una dedizione intensa al proprio mestiere e, dunque, al proprio destino, alla propria ragione di essere di quella cattolicità alla Giuseppe Taliercio, cioè orgogliosa. Presidente, onorevoli colleghi, questa la chiamo virtù. E se un uomo a quella virtù rimane leale e fedele sino in fondo quell'uomo è un eroe!

parlando di testamento biologico, ritengo che coloro che sostengono questa tesi non abbiano voluto davvero affermarla, ma sostanzialmente cercato, come si usa fare da parecchio tempo, di aggirare un problema che, obiettivamente, è avvertito non soltanto in Italia

quando afferma che si mette in discussione il diritto di libertà del cittadino. La questione non è così semplice. Il tema è molto complesso e riguarda lo stesso contenuto della Costituzione. Il quesito che ciascuno di noi deve porsi è proprio che tipo di Costituzione è la nostra. Si vuole affermare qui che questa Costituzione, frutto di un compromesso mirabile in cui il Partito Comunista di Togliatti

Quale posizione trovò accoglienza nel 1947 nella Costituzione dei Padri costituenti che voi, con le vostre tesi, ci accusate oggi di violare? Quale era la posizione? Quella della difesa di un diritto liberale?

stesso negli Stati Uniti d'America, dove c'è un'altra cultura. In tale contesto le disposizioni della giurisprudenza contano, eccome, ma in Italia, senatore Veronesi, non è così. E non lo è grazie alla sinistra che un giorno sì e l'altro pure afferma che i princìpi di cui alla Parte I della Costituzione sono validi,

è inviolabile anche per chi ne è il titolare. Questo è un concetto fondamentale, radicato e vincente nella Costituzione: un diritto inviolabile per tutti.

come deve finire la sua vita. In un testamento, per norma, si decide quello che succede dopo la morte. Ecco perché basterebbe cambiare la Costituzione. Apriamo allora un dibattito autentico, vero, nel Parlamento e nel Paese su questo principio fondamentale. La sua tesi potrà anche risultare vincente, perché no? perché no? Probabilmente ci incamminiamo tutti verso un concetto secondo il quale ognuno può decidere come morire, però bisogna farlo senza aggirare l'ostacolo, bensì affrontando il problema. E il problema i primi a non volerlo affrontare sono quelli del centrosinistra. La ragione è ovvia: verrebbe meno il Partito Democratico. Ma lei, senatore Veronesi, che pensa, che se ci fosse in Italia un partito socialdemocratico o autenticamente di sinistra il problema non verrebbe affrontato?

il diritto a vivere bene. Come lei sa, il diritto alla salute, come tale definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, non è il diritto a vivere, ma il diritto a vivere bene, che è un concetto ben preciso.

il diritto alla salute è fondamentale, questo ha un significato, perché una cosa vuol dire inviolabile, altra cosa vuol dire fondamentale. Sull'inviolabilità l'articolo 2 non prevede eccezioni,

I diritti inviolabili dell'uomo esistono e la Repubblica li riconosce. Non li crea, non li determina, non li costituisce: li riconosce. Il diritto alla vita o il diritto a vivere, come si evince da tutto il dibattito della Costituente, è un diritto inviolabile

dell'articolo 32 disciplina la tutela della salute: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo».

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite (...). Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

una Repubblica che si fa carico, una Repubblica che promuove, una Repubblica che non è assente rispetto ai diritti del cittadino, ma che diventa parte e alleata del cittadino tutela la salute.

cosa c'è di strano nel disegno di legge in esame? Non attua forse questo principio? Questo disegno di legge non consente a ciascuno di noi di rinunciare all'idea di vivere bene, cioè al diritto alla salute, come previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità, come stato di benessere psicofisico?

che questa maggioranza, per un eccesso di apertura nei confronti dell'opposizione, è andata oltre, concedendo molto rispetto ad una Costituzione che è chiara e ben precisa e che nessuno, con riferimento ai princìpi

non sarebbe stato messo all'ordine del giorno, se non fosse accaduto quell'episodio che ha tanto impegnato e scosso l'opinione pubblica nazionale. Intendo riferirmi al caso della giovane Eluana.

Ognuno di noi ha la sua opinione su questa materia ed è giusto che la esprima e che, in funzione del concorso di queste opinioni, si pervenga al risultato migliore, nell'interesse superiore della maggioranza del popolo italiano. Per quanto mi riguarda, quando

dirò subito che il disegno di legge oggi in discussione rappresenta un punto elevato di mediazione o, se vogliamo, un compromesso di qualità tra il diritto all'autodeterminazione della persona e il dovere costituzionale dello Stato di tutelare la vita di ogni singola persona. Difatti, il provvedimento in esame vieta sotto qualunque forma sia l'eutanasia che l'accanimento terapeutico, recependo il principio stabilito dalla mozione approvata dal Senato all'indomani della morte di Eluana Englaro, secondo la quale la nutrizione e l'idratazione, comunque fornite, sono da considerarsi quali forme di sostegno vitale e quindi, come tali, sempre dovute al paziente per ragioni etiche, oltre che deontologiche e giuridiche. Certo, in linea di principio, sarebbe stato meglio non dover legiferare in una sfera come quella del passaggio dalla vita alla morte, onde evitare allo Stato di entrare nell'intimità delle nostre coscienze, dove spesso ci interroghiamo sul mistero dell'esistenza, cercando affannosamente risposte che gelosamente teniamo per noi. Ma diciamoci la verità, colleghi: a questo intervento il legislatore è stato costretto dall'invadenza di campo della magistratura, la quale, profittando del vuoto normativo, ha di fatto regolamentato la materia attraverso sentenze mirate che hanno scandito la breve vita e sancito la tragica morte della povera Eluana. Eluana. Allora, ben venga la legge, questa legge capace di garantire ad ogni cittadino, nel rispetto della sua libertà di scelta, la certezza di cure idonee e di un'adeguata assistenza per la fase terminale dalla sua esistenza, quando magari particolari condizioni psicofisiche non gli consentiranno più di provvedere autonomamente alle proprie fondamentali necessità vitali. Ma la legge, questa legge, si rende necessaria anche per contrastare con la forza del diritto un certo clima culturale che punta a legittimare l'eutanasia, spacciandola addirittura per un semplice diritto di libertà. È un movimento d'impronta nichilista che, utilizzando disinvoltamente gli schemi del relativismo etico, non si ferma di fronte a niente e a nessuno, strumentalizzando persino il dolore delle persone e il ruolo delle istituzioni, come è avvenuto in questi giorni a Firenze, dove il Consiglio comunale ha deliberato a maggioranza di concedere la cittadinanza onoraria a Beppino Englaro, assegnando a tale simbolico atto il senso oggettivo di una condivisione delle ragioni e delle scelte morali del signor Englaro; una forzatura di parte, che ignora il comune sentire di quella città per apportare il suo interessato contributo politico ad una battaglia in favore dell'eutanasia che si fa, purtroppo, sempre più aperta e dichiarata. Ebbene, a questa pericolosa deriva nichilista io non intendo assolutamente rassegnarmi, e lo dico da laico. Da laico che non accetta che il laicismo si trasformi nell'oscena caricatura di un relativismo ridotto oramai a pura espressione di qualunquismo ideologico; da laico che ritiene che la ragione non possa essere mutilata, impedendole di percepire e giudicare i valori morali; da laico che crede che la libertà della propria coscienza sia fondata su valori che la trascendono e la orientano, a cominciare dal valore della sacralità della vita; da laico, insomma, che ritiene che la propria libertà debba farsi responsabilità di fronte alla consapevolezza dell'esistenza di un senso del limite che altro non è, a ben vedere, che il senso del sacro. *(Applausi dal

nei 40 giorni successivi al drammatico confronto svoltosi in quest'Aula, mi sono spesso interrogato su come si sarebbero posti i Padri costituenti di fronte al delicato tema alla nostra attenzione, ovvero come loro avrebbero istruito, affrontato e risolto sul piano legislativo. Sia ben chiaro, si tratta di un interrogativo che non intende assolutamente negare la sovranità di questa nostra Camera, ma che credo può sollecitare in tutti noi un riferimento obbligato a quella straordinaria pagina della nostra vita repubblicana dove culture, filosofie politiche, convincimenti etici e religiosi, seppero incontrarsi su princìpi e valori universali quali la giustizia sociale, la solidarietà, il rispetto della persona umana, la libertà dell'individuo. Come avrebbero trasferito, dunque, in un testo di legge sul testamento biologico e il fine vita il comma 2 dell' articolo 32 della Costituzione, là dove si riconosce che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana? Non si può certo negare che a quella stagione sono seguite molte cose, quali ad esempio lo straordinario sviluppo della scienza, della tecnica, della medicina; la sconfitta storica di un sistema ideologico che in nome della giustizia sociale negava le libertà individuali e la centralità della persona; l'affermarsi nel mondo cristiano, cattolico in particolare, del pensiero del personalismo di Jacques Maritain e del Concilio Vaticano II che tanto hanno illuminato l'azione e le riflessioni di Giovanni XXIII e in particolare di Paolo VI; e, ancora, l'insorgere nel mondo occidentale, a partire dagli Stati Uniti, di una cultura politica, fatta propria dalla destra di quel Paese, al governo per circa due decenni, caratterizzata da un nuovo pensiero di stampo fortemente conservatore tanto da rompere a parere di moltissimi gli ormeggi con gli stessi padri del pensiero liberale, da John Locke a John Stuart Mill, per non parlare dello stesso Kant. Di acqua sotto i ponti dal periodo costituente ne è passata davvero tantissima. Resto convinto in ogni caso che quella eccezionale esperienza, quella ricerca di dialogo e possibile incontro tra diversi umanesimi resti, anche alla luce del presente storico, l'unica bussola in grado di portare ad un saldo ancoraggio la nostra cultura civile e politica. In un recente articolo apparso su un quotidiano nazionale la filosofa Claudia Mancina rilevava, tra l'altro, l'esistenza di una dimensione politica dei temi etici che -cito testualmente - «riguarda l'individuazione dei princìpi sui quali una legge deve fondarsi, princìpi politici che consentano a ciascuno di seguire i propri princìpi etici». Ecco, in tutta la sua profondità, il tema vero al centro della nostra attenzione, al di là di ogni possibile dissertazione intorno alle attuali conquiste della scienza, alle possibili teorie giuridiche o ai filoni di pensiero culturale. La politica, in tutta la sua centralità e autonomia, è chiamata in questa occasione ad essere lo strumento per rendere possibile ogni sforzo, tale da corrispondere all'esigenza di condurre i diversi sentire in un luogo comune condiviso da tutti. Il luogo appunto dove i princìpi politici permettano a ognuno di noi di ritrovare i propri princìpi etici. Il luogo della legge, quindi, riconosciuta come propria da ciascuno e incidente per tutti. Princìpi e, aggiungo, valori condivisi dovrebbero perciò muovere il nostro lavoro proprio su questioni di così grande significato per la vita di ogni persona,

La Carta ci indica i princìpi ed i valori fondamentali a cui è necessario fare riferimento in questo delicato lavoro, a partire dal supremo riconoscimento della libertà dell'individuo. Intervenire su un tema così legato alla dimensione intima di ciascuna persona, quale è il fine vita, non corrispondendo a quel principio fondamentale significherebbe, a mio avviso, non ottemperare al riferimento costituzionale che governa la nostra convivenza democratica. Negando, come nel caso alla nostra attenzione, la libera ed autonoma determinazione dell'individuo si priva la persona umana della sua centralità, collocandola, da un lato, ad acritico strumento del progresso tecnico-scientifico, dall'altro lato, a possibile oggetto dell'inclusione di una autorità pubblica, che si fa Stato etico, non trovando così più limite neppure nell'intima sfera della libertà e della volontà individuale. Il salto sarebbe a mio avviso oltremodo criticabile e pericoloso proprio per il nostro sentire civile e democratico poiché si giungerebbe a trasformare i cittadini in possibili sudditi. Sono perciò dell'avviso che il provvedimento, per come oggi si presenta al nostro esame, sia pericolosamente lontano da quella sintesi tra umanesimi che ha portato i costituenti ad esaltare il valore supremo del rispetto di ogni persona umana. Da qui la mia personale critica al testo in discussione. Negare la libertà di scelta ad una persona sul fine vita o perlomeno fortemente condizionarla appare a mio avviso come un indebito superamento di quei valori e princìpi condivisi che fissano la nostra Carta costituzionale. Non si tratta, certo, di impedire od ostacolare l'obiettivo di un possibile proficuo incontro tra libertà di scelta e tutela della vita, ma ciò va fatto assumendo la piena consapevolezza dell'esistenza di diverse opinioni di merito e nel fondamentale assunto che alla persona umana deve essere riconosciuta la possibilità di decidere sul proprio destino e sulla propria vita. Da qui, il mio personale auspicio che la proposta in discussione possa trovare nel confronto parlamentare un nuovo approdo, una radicale revisione nei contenuti e nelle previsioni affinché si possa trovare efficacemente quella cifra, rispettosa dei limiti imposti al rispetto della persona, della sua libertà, oggi così fortemente condizionati dall'impressionante sviluppo della tecnica e della scienza e tali da incidere, come ricordato in i diversi interventi, perfino sulla naturale conclusione del nostro percorso di vita. Se non risultasse raggiungibile un simile obiettivo, credo si potrebbe determinare uno scostamento di fatto dal disegno sotteso al dettato costituzionale, affermando, al contrario, uno Stato che si sostituisce all'individuo ed alla sua volontà. Una tale eventualità, signor Presidente, certo oggi non così remota, stante il livello del confronto fin qui realizzato, dovrebbe consigliare tutte le parti in causa ad una più attenta riflessione ed analisi degli effetti concreti che si potrebbero determinare. Peraltro, così facendo sì potrebbe perlomeno ascoltare e forse meglio recepire ciò che in grandissima parte lo stesso mondo scientifico e la medicina più avanzata suggeriscono a noi tutti in materia di fine vita e di cure palliative. Di una cosa, signor Presidente, sono quindi persuaso: così avrebbero sicuramente fatto i nostri Costituenti.

credo che dobbiamo inserire in maniera più esplicita questa nostra discussione nel quadro attuale della medicina, della ricerca e delle nuove tecnologie. Molte delle questioni sulle quali il Parlamento è chiamato a legiferare, infatti, sono legate ai progressi della scienza e della tecnica, che hanno sconvolto la naturalità della vita, hanno cambiato le frontiere della nascita e della morte, hanno introdotto elementi di artificialità inimmaginabili fino a non moltissimi anni fa, hanno creato una condizione che sta sospesa tra la vita e la morte. La sopravvivenza molto spesso è legata all'intervento delle macchine anche per la nutrizione; si è stabilito cioè un legame del tutto inedito tra la vita e la tecnica e tra la vita, la tecnica e la politica, chiamata a stabilire regole e leggi: è nata la biopolitica. È il potere politico, cioè, che si fa potere di vita, potere sulla vita dei singoli, un fatto quanto mai illiberale. Quello che non dovrebbe accadere è che lo Stato, grazie a questo legame, imponga una sorta di costrizione a vivere a tutti costi, quali che siano la volontà della persona e le condizioni reali della sua vita, quindi anche uno stato vegetativo persistente per moltissimi anni. Si sancirebbe in questo modo una sorta di obbligo ad essere prigionieri della tecnica. Ad un certo punto, sarebbero le macchine a possedere i nostri corpi e le nostra volontà: le macchine si appropriano della nostra vita, diventiamo proprietà delle macchine. Ma in questo modo si arriva alla negazione della persona umana e della sua dignità, in quanto capace di libera scelta. Non possiamo, come legislatori, sancire questo ed escludere, anche in presenza di un'espressa volontà, la possibilità di sottrarsi alla tecnica e ritornare alla naturalità della morte. Non voglio fare l'antimoderna, ma è evidente che dobbiamo introdurre un limite alla pervasività della tecnica rispetto alla volontà umana, soprattutto quando si tratta del fine vita. Voglio ricordare a questo proposito una riflessione di Paolo VI, tanto più importante in quanto le attuali gerarchie ecclesiastiche sostengono posizioni molto diverse. Diceva Paolo VI nel 1970: «Il carattere sacro della vita è ciò che obbliga il medico a dedicarsi con tutte le risorse della sua arte a lottare contro la morte. Questo non significa, tuttavia, obbligarlo ad utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza che gli offre una scienza instancabilmente creatrice. In molti casi non sarebbe forse un'inutile tortura imporre la rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabile? In quel caso il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza, invece di prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il suo epilogo». Ho trovato, signor Presidente, colleghi, profondamente sbagliata, perché prevaricante nella sua banale semplificazione e persino offensiva, la contrapposizione estrema a cui si è fatto e si continua ancora a fare ricorso fra cultura della vita e cultura della morte. Si tratta invece, dobbiamo accettarlo tutti, di differenti concezioni della vita e della dignità della morte e nella morte. Anche in questo caso, io, non credente, voglio citare le parole sagge, vorrei dire misericordiose, di un prelato, monsignor Casale, vescovo emerito di Foggia, che, durante le polemiche sulla morte di Eluana Englaro, ha rifiutato quell'accusa terribile di assassinio risuonata anche in quest'Aula

Personalmente, ritengo inaccettabile una concezione sacrale della vita che prescinda dalle condizioni concrete dei soggetti e dalla volontà individuale, come se potesse darsi una vita astratta e metafisica. Vorrei porre, invece, al centro della nostra attenzione il valore della dignità della persona umana in tutte le fasi della vita, fino al momento della morte. C'è una dignità umana nel vivere e una dignità umana nella morte. La dignità, per essere e manifestarsi, deve contenere ed esigere forme di rispetto: il rispetto della vita e il rispetto della libertà di ciascuno di decidere come vivere il fine vita. Non vi è dignità senza questa libertà, una libertà costituzionale certamente chiarissima nell'articolo 32 della Costituzione, molte volte citato. Anch'io voglio richiamare quel passaggio che pone limiti alla legge: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Quel rispetto della persona umana implica, contiene, il rispetto della sua volontà, fosse anche quella di rifiutare le cure, una volontà che porta alla morte, per quanto ciò sia doloroso da accettare. La Costituzione ci conferma che l'indisponibilità della vita umana riguarda in primo luogo lo Stato. Una legge sul testamento biologico che non prevedesse la possibilità di rinunciare alla cura e anche alla vita, non sarebbe conforme all'articolo 32 della Costituzione, perché non sarebbe rispettosa della volontà individuale e perché sancirebbe un affidamento della vita individuale allo Stato. È il caso di richiamare un passaggio importante della sentenza della Suprema Corte, che recita: «Il diritto costituzionale di rifiutare le cure è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone *erga omnes*». Dunque, è compito del legislatore arrivare ad approvare un testo sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che preveda tutte le garanzie di rispetto, sia per la vita della persona, che per le sue libere decisioni: due valori costituzionali che vanno tenuti insieme. È qui la sfida del legislatore e mi auguro - anche se i richiami all'ordine che sono arrivati da luoghi apicali del Governo lo lascerebbero escludere - che in quest'Aula si creino le condizioni di ascolto anche delle nostre ragioni, le ragioni cioè di chi non ritiene che si possa affermare la dignità della persona umana se le si nega la possibilità di decidere del suo fine vita. Considero l'ascolto delle ragioni che ciascuno porta nella discussione tanto più necessario, in quanto sono sempre più convinta che leggi su materie così sensibili, che chiamano in causa coscienza individuale e convincimenti etici e religiosi, debbano essere in grado di rispecchiare i diversi punti di vista e la molteplicità delle posizioni etiche che esistono nella società. che vanno rispettate, lo voglio dire al senatore Nania, e non irrise come lui ha fatto con molta supponenza e arroganza. È questo il compito dello Stato laico, che agisce in autonomia, con l'unico scopo di costruire il bene comune. La storia parlamentare della nostra Repubblica, con le riforme degli anni '70 e '90, rivelatesi sagge e lungimiranti, dimostra che questo è possibile e lo è tanto più se si tiene ferma la centralità del Parlamento. Vorremmo che ciò accadesse anche in questo caso. Nei giorni scorsi è stato ripetuto molte volte che ci stiamo occupando di questioni sulle quali nessuno possiede la verità. È giusto. Tanto più, allora, la politica non ha il compito di cercare o affermare la verità, ma è chiamata a fare pratica di ragionevolezza, a cercare punti di convergenza e di mediazione. Solo la ragionevolezza ci consente infatti di tenere conto del pluralismo e delle molteplici posizioni etiche che si confrontano. Certo, nella democrazia alla fine è una maggioranza che decide, ma il risultato sarà tanto più convincente e condiviso quanto più il processo che porta alla decisione ha visto un confronto aperto e libero e non una volontà di prevaricazione e di chiusura. Mi piacerebbe poter fare riferimento a una sorta di etica del legislatore, ispirata alla responsabilità. Non che i princìpi non siano importanti, anzi. È però la responsabilità che ci costringe a farci carico delle ragioni dell'altro, a tenere conto del pluralismo esistente, a esercitare l'autonomia della politica e a rispondere non solo alla propria coscienza, ma anche ai destinatari della legge. Ognuno porta nella discussione i suoi valori e i suoi princìpi, ma alla fine il risultato, il prodotto, dovrebbe essere una proposta che riesca a tenere insieme almeno le posizioni maggiormente condivise. In Commissione qualcosa à accaduto. Rispetto a un testo che stravolgeva completamente la Costituzione, qualche correzione è stata fatta, ma per noi sono cambiamenti insufficienti. Restano ancora diversi punti che ci fanno dare un parere negativo e dei quali hanno parlato altri colleghi, tra cui i senatori Veronesi e Marino. Voglio Voglio richiamare il tema per me centrale, ossia l'impossibilità di inserire nella dichiarazione anticipata di trattamento l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione. È un ragionamento di buon senso sostenere che come il paziente cosciente ha il diritto di rifiutare di essere alimentato con il sondino, così questo deve poter essere staccato anche a quello incosciente, quando ciò corrisponda alla sua volontà. Ciò viene invece negato nel testo in discussione. Noi vogliamo offrire - questa è una riflessione politica che ritengo importante - all'attenzione dell'Aula la proposta che il Gruppo del Partito Democratico ha elaborato in una lunga e profonda riflessione, in una discussione che si è svolta alla luce del sole, su un punto controverso come quello che ho citato. Come risulta anche dagli emendamenti che abbiamo presentato - voglio citare i particolare quello di cui è prima firmataria la senatrice Finocchiaro - si prevede che alimentazione e idratazione siano sempre garantite, salvo che non vi sia una diversa volontà espressamente dichiarata dalla persona. Vengono in questo modo salvaguardate garanzie di sopravvivenza e possibilità di espressione di una volontà liberamente dichiarata e rispettata, che per la nostra Costituzione è incomprimibile.

che ci apprestiamo a varare è certamente una legge difficile da fare e credo ancora più difficile da spiegare, qualunque essa sia, perché affronta un tema di assoluta rilevanza per ogni sistema parlamentare e per ogni persona. Vi giungiamo, tra l'altro, con i postumi di uno strappo nella coscienza e nell'esperienza del nostro popolo, costituito dall'uccisione di Eluana Englaro. Speriamo però che tutto ciò non sia accaduto invano,

Era ormai inevitabile legiferare su questo tema, ma occorre dire, prima di scegliere e votare, che questa legge comunque introduce nel nostro ordinamento princìpi assolutamente innovativi in tema di tutela e difesa della vita, come mai era accaduto prima. La necessità di porre ordine in tale materia non può però farci dimenticare che tipo di *vulnus* si introduce nel nostro sistema e molto di più nella nostra convivenza sociale; posso affermare ciò perché sono un convinto assertore della difesa del valore della vita senza se e senza ma, dal concepimento alla morte. morte. Con questa legge, invece, si introdurranno comunque possibilità, e speriamo che ciò non accada, che possono aprire all'utilizzo dell'eutanasia, principio e metodo che abbiamo sempre rifiutato e contro cui ci batteremo. Ricordo che presi particolare coscienza di questa drammaticità quando, all'inizio della discussione sul caso Englaro, una sera ascoltai un dibattito televisivo cui seguì un altro programma, un servizio sull'antica Grecia. Si illustrò la differenza tra la civiltà di Atene e quella di Sparta, fino a descrivere - come tutti ricordiamo dai libri di scuola - la selezione che si faceva a Sparta dei bambini appena nati. La nostra odierna società è certamente più complessa e sofisticata, e quindi utilizza sistemi meno grossolani, ma forse il desiderio di intervenire anche sulla qualità del genere umano potrà avvenire. È per questo che il dibattito in Parlamento e nel Paese deve essere sì pacato, ma anche approfondito e in grado di cogliere tutte le connessioni. C'è il rischio, Presidente, che mentre a Roma si tenta di introdurre larvati princìpi sull'eutanasia, a Modica, in Sicilia, di fronte ad un branco di cani che ha fatto - speriamo - una sola vittima, c'è che sostiene che, pur nell'emergenza, i cani non debbano essere abbattuti, ma solamente catturati. Occorre necessariamente partire dalla perdita del significato della sofferenza: essa è un antico nemico con cui l'umanità ha sempre dovuto fare i conti, ma acquista un volto particolarmente spaventoso in una cultura come la nostra, dove il valore fondamentale è diventato quello della piena realizzazione delle proprie facoltà e delle proprie aspirazioni. anche l'eutanasia diventa una soluzione inevitabile ed auspicabile di una vita ritenuta inutile o addirittura dannosa, un male da estirpare. La qualità della vita è uno dei sentimenti che porta alla domanda di eutanasia, anche se spesso non è il sentimento del malato, ma quello di chi segue il malato, di chi non riesce a sopportare lo sguardo di chi vuole aiuto, di chi domanda il perché della sua condizione. Diventano domande da sopprimere piuttosto che da affrontare. Eppure, a ben vedere, proprio l'incontrastato dominio di questo modo di intendere la vita rischia di oscurare qualcosa di essenziale, che forse proprio la sofferenza potrebbe portare alla luce. Questo qualcosa è la stessa realtà dell'io. Nel rapporto con la sofferenza vengono fuori le domande ultime dell'uomo. In realtà, tutta la cultura oggi dominante risale a maestri che hanno rigorosamente negato la realtà del soggetto. Per Nietzsche, come poi per Freud, non è l'io consapevole il centro della realtà dell'uomo: Nietzsche parla di un caos perennemente fluente e inafferrabile, di cui la cosiddetta coscienza è soltanto una maschera semplificata, artificialmente sovrapposta per motivi pratici; Freud privilegia la sfera dell'*es* - terza persona singolare neutra, dunque qualcosa non qualcuno - che si identifica con l'inconscio. Entrambe le teorie convergono nel denunziare l'artificiosità e il carattere solo strumentale e sostanzialmente repressivo della sfera conscia dell'uomo. Quello che un tempo si considerava il centro della persona, su cui misurare il suo essere e il suo agire, l'anima, è diventato, così, un concetto da museo. La malattia ci mette nudi di fronte alla realtà; non possiamo drogarci, come facciamo usualmente per affrontare la quotidianità, come spesso siamo costretti per vivere al *top*. Si parla tanto di vite sprecate - scrive ancora Kierkegaard - ma sprecata è soltanto la vita di quell'uomo che così la lasciava passare, ingannato dalle gioie della vita e dalle preoccupazioni, in modo che non diventò mai, con una decisione eterna, consapevole di se stesso come spirito, come «io». Certo, ciò non è automatico, la sofferenza può anche distruggere o incattivire. L'uomo, la donna che soffrono si sentono incompresi da tutti, si sentono un peso per tutti. La sofferenza, inoltre, può dare un senso di credito verso la vita e verso gli altri. Perciò, nella sofferenza, davanti allo spettacolo della propria decadenza decadenza fisica e psichica, si può diventare meno persone. Ma è possibile anche un processo diverso, sebbene certamente non privo di drammaticità e sicuramente irriducibile ad ogni retorica del dolore che rende migliori. La sofferenza e la malattia possono produrre una disperazione che, facendo crollare il falso io e aprendo lo spazio a quello autentico, costituisce l'antidoto a quella disperazione più sottile che si nasconde dietro il mito del superuomo. Il perno della giustificazione che si vuole accampare e far valere di fronte all'opinione pubblica è sostanzialmente costituito da due idee fondamentali: da un lato dal principio di autonomia del soggetto, il quale avrebbe diritto di disporre in maniera assoluta della propria vita; dalla persuasione dell'indebolimento spirituale e morale riguardo alla dignità della persona morente e una via utilitarista di disimpegno di fronte alle vere necessità del paziente, più o meno esplicitate, legate all'insopportabilità e inutilità del dolore che può talora accompagnare la morte. L'esperienza degli *hospice*, cliniche il cui obiettivo primario è l'umanizzazione dell'assistenza ai pazienti in fin di vita, e il trattamento del dolore - attraverso le cosiddette cure palliative - mette in dubbio ulteriormente la correlazione fra sofferenza e desiderio di morire,

In ogni caso, la sofferenza non è solitamente un fattore di rischio indipendente. La variabile significativa nel rapporto fra sofferenza e suicidio è l'interazione fra sofferenza e sentimenti di disperazione e depressione. Questo lungo ragionamento è necessario per assumere posizione sulla questione più controversa: l'alimentazione e l'idratazione. Un cedimento su questo terreno, come è avvenuto nel caso della morte di Eluana, apre necessariamente ad altro, ad un arbitrio dell'uomo, chiamato magari libertà o autodeterminazione, di cui non si è in grado di prevedere dove possa condurre. testé richiamate ci inducono a sostenere un disegno di legge, la cui mancata approvazione potrebbe dare luogo ad una giungla peggiore di quella in cui ci troviamo, nella quale giudici e strumenti amministrativi hanno la prevalenza sul comune sentire e sulla difesa di valori fondanti la nostra convivenza.

che ci impone di approvare una legge che sia il frutto di un libero confronto tra diverse sensibilità politiche, etiche e religiose e non la schematica trasposizione giuridica delle tesi cattoliche sulla vita e sulla morte. Analogamente credo che tutto le confessioni religiose si debbano astenere dall'ingerirsi nelle decisioni prese dai diversi poteri di uno Stato laico, come quello italiano, e che in materia di coscienza e di fede nessuno possa imporre con la coercizione convinzioni ispirate a qualsiasi credo. Per questo auspico un confronto davvero pluralistico e non affrettato su un tema così delicato. La laicità, dunque, quale valore irrinunciabile di uno Stato, in quanto valore irrinunciabile della nostra Carta costituzionale. Laicità significa che nessuna convinzione religiosa o morale viene imposta per legge da un gruppo di persone, per quanto ampio, alla totalità dei cittadini. Ed allora possiamo serenamente partire da alcuni princìpi faro, sono stati già richiamati negli interventi di questa mattina. La Costituzione della Repubblica nel suo articolo 32, la Convenzione di Oviedo e numerose sentenze della Cassazione degli ultimi anni stabiliscono in modo tassativo che nessun cittadino - ripeto nessun cittadino - può essere sottomesso a interventi nel campo della salute senza il suo consenso (debitamente informato) e che tale consenso può essere ritirato in qualsiasi momento. La Convenzione di Oviedo poi evita ogni distinzione tra cura e altri interventi di sostegno vitale, proprio perché non si possa giocare sulle parole e violare così il diritto del paziente a rifiutare un trattamento medico-ospedaliero (tranne che ovviamente nei casi eccezionali di epidemie, vaccini e per motivi di sicurezza pubblica). Allora Allora cosa si può e si deve fare per accordare il diritto positivo alle emergenze valoriali dell'etica di fine vita indotte dal progresso tecnologico in medicina, che oggi ci dà possibilità d'intervento e di omissione nella cura prima impensabili? La buona pratica medica sa che i protocolli scientifici e terapeutici sono sempre da interpretare al letto del malato, che è una persona concreta, un'individualità effettiva anche come risposta meramente biologica alle terapie e non un caso clinico come semplice ricorrenza statistica di una fenomenologia patologica, affrontabile sempre e comunque nello stesso modo. In questo settore, dove niente è pacifico, dove lo stato vegetativo permanente non trova nel criterio della morte cerebrale un'univoca percezione che con l'integrità della persona sia anche cessata l'individualità non disponibile della sua vita biologica, che non è un cadavere ma che non è neanche certo più una persona, che fare? I valori che entrano in conflitto sono noti. Da un lato c'è l'evidenza ontologica dell'indisponibilità individuale della vita, dall'altro c'è il valore dell'autonomia individuale la cui scoperta e la cui enfasi ha storicamente costruito la possibilità stessa dei diritti umani. Come rispettare quella evidenza senza ledere questo valore? L'unica strada percorribile è forse attenersi proprio al lascito personale di una volontà espressa nella pienezza dell'autonomia della persona; da qui la liceità e l'importanza delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Se l'individuo con diagnosi di stato vegetativo permanente, irreversibile secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, abbia nella pienezza della sua autonomia di persona espresso la volontà di non ricevere sostegni terapeutici alla sua vita biologica quando sia venuta meno in modo irreversibile ogni possibilità di restituirlo al suo stato di persona e non accetti di non poter esser più persona, qualunque cosa sia nell'interregno che lo separa dallo stato certo di cadavere, una vita in stato vegetativo permanente con perdita delle funzioni della corteccia cerebrale rigorosamente accertata, dove è venuta meno l'integrazione psicofisica alla base della possibilità stessa della vita cosciente, credo sia una vita che può ben essere accompagnata a spegnersi, lasciandola al corso naturale delle cose senza accanimento terapeutico. Lo slittamento semantico da testamento a dichiarazione anticipata di trattamento non credo sia neutro; tende a depotenziare il carattere rigidamente vincolante di una disposizione testamentaria. Quello che si vuole, credo, con questo slittamento semantico è, in definitiva, uno stato interpretativo aperto delle decisioni di fine vita che trovi la sua concreta definizione al letto del malato, lì effettivamente ascoltato nelle sue volontà disposte; che, in altri termini, quelle decisioni non discendano *sic et sempliciter* da una disposizione testamentaria ora per allora, che può farsi anche obsoleta alla luce dei progressi della medicina. Ora, però, proprio questa giusta esigenza, che la norma garantisca uno stato interpretativo aperto, affidato all'alleanza terapeutica tra medico e paziente (ovvero il fiduciario che lo rappresenta) nelle cure di fino vita, non può tradursi nella non assimilazione a priori dell'idratazione e dell'alimentazione all'accanimento terapeutico. L'esclusione a priori, infatti, dell'idratazione e dell'alimentazione quali terapie, decidendo anticipatamente per legge che non costituiscono in nessun caso terapia e, dunque, neppure accanimento terapeutico, chiuderebbe di fatto lo stato interpretativo aperto di un'alleanza terapeutica che si senta impegnata ad ascoltare nella situazione effettiva il paziente. infatti, che l'accanimento non sia semplicemente configurato dal ricorso o dall'esclusione di questa o quella tecnica, ma sia il complesso di un approccio finalizzato della cura che ha perso la proporzionalità tra mezzi e fini.

In tal modo, con questa norma così come è scritta, la dichiarazione anticipata di trattamento diventa una beffa. Qualsiasi cosa abbia deciso un nostro concittadino in alleanza terapeutica con il medico, qualunque sia la sua volontà, lo vedremmo costretto a a recepire un sondino che gli verrà messo in gola a forza. Ho già detto che questa è, ovviamente, la questione centrale, o comunque una delle principali, di questo disegno Ed è su questo punto che auspico si realizzi il massimo sforzo per venire incontro a tutte quelle esigenze plurali richiamate all'inizio del mio intervento, affinché si possa individuare una soluzione che ci consenta serenamente di affermare

*(PD)*. Signor Presidente, vorrei muovere qualche considerazione partendo dalle conclusioni dell'intervento della collega la quale in maniera molto efficace ha voluto offrirci una chiave interpretativa, che purtroppo risulta alquanto originale, sull'espressione laicità e su cosa sia la laicità. Questo non solo perché molte volte è capitato nel passato, ma anche nella nostra età contemporanea, che il concetto di laicità sia stato associato a quello di laicismo, ma perché c'è bisogno di scovare di quest'espressione non soltanto l'aspetto etimologico, ma anche quello storico. Fondamentalmente, signor Presidente, se vogliamo cercare di essere semplici, essere laici vuol dire essere portatori sani di dubbi. Essere laici significa essere talvolta tormentati, significa essere privi di quelle certezze granitiche che, a seconda di come vengono declinate, possono indurre all'integralismo o al radicalismo, e possono indurre all'intolleranza e alla mancata accettazione degli altri. Un esempio di questa intolleranza gabellata con una una lezione di diritto costituzionale l'abbiamo avuta anche stamattina quando, in maniera spavalda, il senatore Nania ha ritenuto di doverci apostrofare, mirando per primo al senatore Veronesi, per non essere fedeli interpreti del dettato costituzionale. Già questo atteggiamento di per sé rischia di sconfinare nell'autoritarismo e diventa tanto più urticante ed insostenibile quando, muovendo da certe considerazioni, si ha la pretesa di dare la patente agli altri, tanto da definirli, come arditamente il senatore Nania ha fatto, soggetti che da questa parte operano nell'errore. Vorrei sottolineare ulteriormente questo aspetto. Come diceva Carlo Bo di se stesso, io sono soltanto un aspirante cristiano o, se debbo mutuare da un famoso libro di Ignazio Silone, la mia è l'avventura di un povero cristiano. Però desidero proclamare questa mia condizione con molta serenità, senza chiamare con aggettivazioni improponibili in un contesto democratico quanti la pensano diversamente da me, ma senza neppure assumere un atteggiamento di rinuncia rispetto a quanti, proprio in quest'Aula, hanno ritenuto in qualche modo di doverci definire, similmente a quanto fa il supremo (quello che si scrive però con la esse minuscola,

Fatta questa precisazione, sempre da aspirante cristiano, vorrei fare qualche riferimento affinché sia chiaro da questa parte del Tevere, per quanti avessero la ventura di seguirci anche dall'altra parte del Tevere, che noi del Partito Democratico non siamo mossi da nessuna pulsione radicaleggiante (e con questo non intendo naturalmente in alcun modo offendere i miei colleghi radicali, verso i quali verso i quali porto rispetto e dei quali mi onoro di essere compagno di viaggio), però questo è il sistema. Chi non fa parte dell'idea forte secondo cui la vita andrebbe difesa a tutti i costi, è una sorta di assassino *in fieri*, è una sorta di scomunicando, qualcosa comunque di moralmente detestabile. Allora, signor Presidente, rinfrancato dalla sua attenzione e da quella dei pochi colleghi reduci, vorrei ricordare un'espressione che nel 1970 il grandissimo Paolo VI volle esprimere all'interno di una lettera che indirizzò ai medici. In questa lettera si sosteneva che «il medico non è obbligato ad utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza che gli offre una scienza instancabilmente creatrice. In molti casi non sarebbe forse un'inutile tortura imporre la rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabile?». Poi soggiungeva il grande Paolo VI: «In quel caso il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza invece di voler prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo in qualsiasi condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il suo epilogo». Non mi pare, signor Presidente e cari colleghi, che il Sommo Pontefice, che naturalmente ci rappresenta tutti, rappresenta tutti i credenti, anche la mia modesta persona, abbia mai chiesto perdono all'umanità, così come Papa Giovanni Paolo II ha fatto generosamente per tante volte; non mi pare abbia mai chiesto perdono all'umanità per le dichiarazioni di papa Paolo VI. Non mi pare, cioè, che questa dottrina così esplicita e così chiara sia mai stata confutata da una Chiesa che ha, non solo il diritto, ma anche il dovere di di esprimere la propria opinione riguardo gli accadimenti dell'umanità e quindi anche del nostro Paese. Spetta a noi, come credenti, comunque come credenti laici, dare il giusto posto ai postulati della Chiesa, senza mai perdere di vista il fatto che la nostra Carta,

un altro passaggio di una persona straordinaria, che stimo molto, ossia Enzo Bianchi,il priore della comunità monastica di Bose, il quale ricorda: quanti monaci, quante donne e uomini santi, di fronte alla morte, hanno chiesto di restare soli e di cibarsi solo dell'Eucaristia? Quanti hanno recitato il «*Nunc dimittis*» come ultima preghiera nell'attesa dell'incontro con Colui che hanno tanto cercato? Tra questi, non casualmente, il priore Bianchi cita anche Giovanni Paolo II. E lo cita a ragion veduta, non con un atteggiamento occhiuto, non con un desiderio di strumentalità, non con un cinico calcolo, così com'è accaduto in questa circostanza allorché, per parlare della vita umana di una povera ragazza che stava per lasciare questa vita, si è detto che ci si voleva accanire, che la si voleva tormentare, che la si voleva violare nella sua libertà, ribaltando paradossalmente il termine dei rapporti. Ecco, io mi auguro, signor Presidente e illustri colleghi, che quando dovessimo scandagliare il nostro dettato costituzionale non ci ricordassimo, come ha fatto stamattina - ahinoi! - il maniera alquanto confusa il senatore Nania, solo dell'articolo 2 2 o anche, con lo stesso atteggiamento, dell'articolo 32, ma ci si ricordasse che esiste anche un articolo 3 della Costituzione, un articolo che si fa cura dell'uomo in tutta la sua integrità. È l'articolo dell'umanesimo integrale, è l'articolo dell'amore verso l'uomo come creatura, indipendentemente dalla fede di cui può essere portatore. Allora ci accorgeremmo che difesa della vita non vuol dire soltanto difesa dei diritti e delle prerogative di un morente o di una morente ma anche di chi ha bisogno di essere liberato dal bisogno, ha bisogno di essere inserito in una comunità giusta, ha bisogno di godere di tutti i diritti che sono riconosciuti agli italiani così come per l'appunto l'articolo 3 stabilisce.

Signor Presidente, signor relatore, signor rappresentante del Governo, colleghi, da persona che ha cominciato da meno di un anno la propria esperienza politica sento forse più di altri di vivere un momento importante per il nostro Paese. Sono chiamato a pronunciarmi, però, su un tema di cui ignoro gli aspetti tecnici ed, essendo di professione un ricercatore, affronto l'argomento studiando e ascoltando quelli che sanno, cioè i medici in primo luogo e i costituzionalisti. Ho letto e ascoltato posizioni scientificamente contrastanti, talora addirittura contrapposte, molte delle quali autorevolmente e credibilmente documentate. Allora devo fare ricorso, più che alla tecnica, alla mia sensibilità che però forse, per gli aspetti che dicevo, potrebbe essere meno lontana da quella comune rispetto a quella di chi si trova da molti anni in quest'Aula. La mia sensibilità mi dice prima di tutto che è giusto che una legge ci sia, di fronte all'effetto collaterale che lo straordinario progresso della scienza medica sta producendo. L'assenza di una legge ha, per esempio, prodotto quella traballante, a mio avviso, volontaria giurisdizione del caso Englaro che sostituiva, appunto, una funzione legislativa tuttora e fino a quel momento carente. Per altro verso sono del tutto contrario a certe zone grigie teorizzate da alcuni che richiedono un'alta capacità dei medici e un contesto di amore familiare che, di questi tempi, rischia di essere l'eccezione più che la norma. Quanto al giudizio politico, io credo e continuo a credere nella libertà individuale, temperata dal superiore interesse collettivo in misura residuale ove esista un interesse collettivo. Credo dunque nella libertà di ciascuno di scegliere secondo i propri valori, la propria coscienza, ed eventualmente la propria fede a quali condizioni vivere e a quali condizioni morire. In questo mi spingo forse lontano da tutte o quasi le diverse visioni del problema che in quest'Aula sono state espresse, che hanno dato luogo alla presentazione Non mi sfugge il confine della libertà individuale, che è - ed è giusto che sia - quello oltre il quale si lede il diritto di qualcun altro o addirittura si lede il bene della comunità a cui l'individuo appartiene. Ma in effetti che cosa viene qui leso? L'interesse alla buona salute di un'intera comunità è sì un interesse collettivo, perché tende a salvaguardare i rapporti sociali e persino quelli economici, ma la posizione dei singoli individui, nell'alternativa tra la vita vegetativa e la morte, collettivo. *(Applausi del senatore Perduca)*. La sopravvivenza in queste condizioni non giova alla collettività più di quanto possa nuocere al malato che non la desideri e persino, scusate il cinismo, dal punto di vista della migliore destinazione delle limitate risorse della sanità pubblica. La tutela della salute è un diritto dell'individuo e non un interesse collettivo e la libertà individuale è una delle radici della società europea, almeno quanto il patrimonio dei valori cristiani, che peraltro non verrebbero certo disconosciuti, permanesse la libertà di ciascuno di vedere tutelato il proprio diritto a vivere o a sopravvivere, anche in condizioni estreme. Ma si tratta appunto di un diritto e non di un dovere. In questa posizione ha pesato - non vi nascondo - anche una dolorosa esperienza personale. Non auguro a nessuno di coloro che voteranno a favore di questo disegno di legge di dover assistere una persona cara che affronta il progressivo degrado del corpo, della mente e della dignità di fronte a una malattia incurabile. Ma il punto è un altro, dicevamo. Abbiamo il diritto o il dovere di vivere? Abbiamo noi il diritto inviolabile alla vita o altri il diritto di obbligarci a vivere in qualunque condizione? Io personalmente sento il dovere di vivere, ma sento anche che non ho il diritto di imporre questa mia visione agli altri. Allora, credo che purtroppo non potrò votare questo disegno di legge, anche se in astratto ciò dipende da se e come verrà emendato. Ma proprio per questo, consentitemi in conclusione di esprimere il mio forte disagio, da persona un po' nuova all'esperienza politica, rispetto alle tante, troppe strumentalizzazioni politiche cui ho assistito dentro quest'Aula e nel Paese, persino con incredulità.

Credo che questo argomento dovesse essere affrontato dal Parlamento con preciso riferimento alla coscienza individuale, morale e politica di ciascun rappresentante dei cittadini e non con lo scontro fra le parti. Ringrazio ci tengo a farlo - il vertice del mio Gruppo e il *leader* del Popolo della Libertà Silvio Berlusconi, che ancora ieri ha ribadito la libertà di coscienza in materia, con il limite (che condivido, come appunto dimostro con questo intervento) di dichiarare apertamente il proprio orientamento, con responsabilità, senza imboscate sui voti segreti. Proprio Proprio per questo, per evitare ulteriori strumentalizzazioni, non voterò contro il disegno di legge e non mi asterrò, poiché questo al Senato produce effetti equivalenti. Farò invece tutto il possibile per migliorare

Sono costretta a farlo ora, in questo luogo, per evidenziare l'impossibilità di fare altrettanto dopo l'entrata in vigore di questa legge, ma mi costa fatica, molta fatica. Aderisco all'appello lanciato dall'Associazione Luca Coscioni e dall'associazione «A Buon Diritto» di fare in Aula le proprie dichiarazioni anticipate di volontà. Ieri mi ha preceduto il senatore Marco Perduca, ha utilizzato un modello che è a disposizione sul sito Internet dell'Associazione Luca Coscioni. Io utilizzerò un altro modello - proprio per evidenziare che le modalità per fare le dichiarazioni anticipate di volontà sono attualmente

«Io sottoscritta Donatella Poretti, nata ad Arezzo il 14 febbraio 1968 e residente a Firenze, nel pieno delle mie facoltà mentali e allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona, affermo solennemente con questo documento, che deve essere considerato come una vera e propria dichiarazione di volontà, il mio diritto, in caso di malattia, di scegliere tra le diverse possibilità di cura disponibili e al caso anche di rifiutarle tutte, nel rispetto dei miei princìpi e delle scelte di seguito indicate. Intendo inoltre che le dichiarazioni contenute in questo documento abbiano valore anche nell'ipotesi in cui in futuro mi accada di perdere la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni ai miei medici curanti sulle scelte da fare riguardo ad una malattia. A questi fini, prevedo la nomina di un fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà e, se necessario, a sostituirsi a me in tutte le decisioni, affinché queste siano vincolanti per i medici. Considero prive di valore e lesive della mia dignità di persona tutte le situazioni in cui non fossi capace di un'esistenza razionale e/o fossi impossibilitata da una malattia irreversibile a condurre una vita di relazioni e quindi considero non dignitose tutte le situazioni in cui le cure mediche non avessero altro scopo che quello di un mero prolungamento della vita vegetativa. Perciò, dato che in tali circostanze la vita sarebbe per me molto peggiore della morte, voglio che tutti i trattamenti destinati a protrarla siano sospesi o cessati. Considero egualmente non accettabili, in quanto anch'esse peggiori della morte e in contrasto con il mio concetto di valore della vita e dignità della persona umana, situazioni in cui malattie senza prospettive di guarigione siano inutilmente inutilmente prolungate attraverso cure e metodi artificiali. Per questi motivi, dispongo quanto segue: che interventi oggi comunemente definiti "provvedimenti di sostegno vitale" e che consistono in misure urgenti quali, ad esempio, la rianimazione cardiopolmonare, la ventilazione assistita, la dialisi, la chirurgia d'urgenza, le trasfusioni di sangue, l'alimentazione artificiale, terapie antibiotiche, non siano messi in atto qualora il loro risultato fosse, a giudizio di due medici dei quali uno specialista, il prolungamento del mio morire, il mantenimento di uno stato d'incoscienza permanente, il mantenimento di uno stato di demenza, la totale paralisi con incapacità a comunicare. In particolare, nel caso io fossi affetta da una malattia allo stadio terminale, da una malattia o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, da una malattia implicante l'utilizzo permanente di macchine o altri sistemi artificiali, inclusa ogni forma di alimentazione artificiale, e tale da impedirmi una normale vita di relazione, rifiuto qualsiasi forma di rianimazione o continuazione dell'esistenza dipendente da macchine e non voglio più essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico. Chiedo inoltre, formalmente, nel caso fossi affetta da una delle malattie sopraindicate, che siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso in particolare l'uso di farmaci oppiacei, anche se essi rischiassero di anticipare la fine della mia vita. Nella prospettiva, inoltre, di una auspicata depenalizzazione anche nel nostro Paese dell'eutanasia, nel caso in cui anche la sospensione di ogni trattamento terapeutico non determini la morte, chiedo che mi sia praticato il trattamento eutanasico, nel modo che sarà ritenuto più opportuno per la conclusione serena della mia esistenza. disposizioni particolari: non voglio l'assistenza religiosa. Il mio corpo può essere donato per trapianti, il mio corpo può essere utilizzato per scopi scientifici e didattici. Voglio essere cremata. Non voglio funerali o altre cerimonie funebri. Voglio che le mie ceneri vengano disperse nella natura. Ai fini dell'attuazione delle volontà espresse nel presente documento, nomino mio rappresentante fiduciario Marco Perduca, nato a Firenze il 28 aprile 1967 e residente a Firenze. Chiamo a testimonianza di questo presente atto il Governo, i senatori, i funzionari d'Aula e anche il presidente dei Radicali italiani, onorevole Bruno Mellano, che ci assiste dalla tribuna. Deposito la presente dichiarazione ai fiduciari ed ai testimoni sopraindicati. Roma, 19 marzo 2009». 2009». Questa premessa, ripeto, mi costa fatica perché solitamente cerco sempre di intervenire con leggerezza, cercando di alleviare la pesantezza di queste giornate che ci hanno visto confrontare in Commissione. Purtroppo, la costrizione a fare e a leggere questo atto è stata determinata dalle circostanze che temo ci porteranno ad approvare una legge che renderà impossibile che qualcuno possa fare una dichiarazione anticipata di trattamento con queste modalità, con queste indicazioni e nel rispetto di questa legge che stiamo andando a discutere e a votare. Allora, dobbiamo chiederci perché stiamo facendo una legge.

A me piace molto la frase di Goya «il sonno della ragione produce mostri». L'irrazionalità può sposare la fede, ma non può sposare la scienza e non può essere a fondamento di una legge di uno Stato laico. Allora, perché questa legge è mostruosa? È mostruosa da un punto di vista scientifico e anche giuridico: scientifico per quel passaggio davvero mostruoso sull'alimentazione e l'idratazione. La nutrizione artificiale è un complesso di procedure, mediante le quali è possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali di pazienti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale. Si differenzia nutrizione parenterale ci sono dei preparati dell'industria farmaceutica, adeguatamente miscelati, somministrati direttamente nella circolazione sanguigna, attraverso una vena periferica o una vena centrale di grosso calibro mediante l'impiego di cannule o cateteri venosi; quella enterale i nutrienti (naturali o a preparazione industriale) sono somministrati direttamente nella via digestiva a livello dello stomaco, del duodeno o del digiuno, mediante l'impiego di apposite sonde inserite dal naso, dalla bocca o attraverso stomie confezionate all'uopo. La nutrizione artificiale è da considerarsi, a tutti gli effetti, un trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo. non è una misura ordinaria di assistenza, come lavare o imboccare il malato non autosufficiente. Come tutti i trattamenti medici la nutrizione artificiale ha indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati. L'attuazione della nutrizione artificiale prevede il consenso informato del malato o del suo delegato, secondo le norme del codice deontologico. che ho richiamato è della Società italiana di nutrizione parenterale e enterale. Questa è la scienza. La legge dice tutt'altra cosa, è un mostro scientifico quello che prevediamo nella legge. Poi c'è il mostro giuridico: l'indisponibilità della vita. Ma l'indisponibilità della vita che cos'è? Il diritto alla vita è il diritto a vivere o il dovere, l'obbligo di vivere?

la vita sarebbe indisponibile per me, ma diventerebbe disponibile, a disposizione del medico, che anzi sarebbe obbligato a curarmi anche contro i suoi princìpi, secondo la sua scienza e la sua coscienza. Se ne potrebbe davvero parlare molto di questo dovere di vivere, contrario ai diritti umani fondamentali, sanciti dalle carte internazionali, come la Convenzione di Oviedo, come tutte le convenzioni internazionali. Voi addirittura citate, davvero a sproposito, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ma l'avete letta? L'abbiamo persino ratificata nei giorni scorsi. recita, all'articolo 25 (Salute): «Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità

della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata».

non disabili (appunto i capaci e i non capaci di esprimersi), lo stesso diritto, la stessa possibilità di esprimere quel consenso informato. Invece, in questa legge si crea tale disparità. Il consenso informato può essere espresso e può essere richiesto ed è vincolante per il medico e per la persona capace; per l'incapace no, per l'incapace ci dispiace. L'incapace sarà costretto a subire trattamenti sanitari obbligatori. Perché? Perché è incapace.

È ostruzionismo? Oppure è l'uso del Regolamento con rigore e rispetto, per offrire l'opportunità a tutti i senatori di questa Aula,

in un modo terribile in quella Commissione e ne è uscito leggermente migliorato, grazie all'utilizzo del Regolamento, grazie ai tanti interventi dei moltissimi senatori dei moltissimi senatori del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, ma anche di alcuni senatori della maggioranza (pochi, però qualcuno c'è stato), che hanno richiamato tutti alla razionalità e alla necessità di fare un testo utile per i cittadini.

all'inutilità (alla fine forse questo può essere il dato più positivo) della dichiarazione anticipata di trattamento, perché non vincola i medici.

che dipendono dal consenso informato e quindi li impone ad alcuni soggetti, senza la possibilità che questi esprimano un consenso; non chiarisce la soluzione delle controversie peggio, impone il ruolo del medico paternalista, anzi lo reintroduce. decenni, forse centinaia d'anni, che non si vedeva più il medico - e addirittura, grazie a questa legge, lo Stato Stato - acquisire la disponibilità dei corpi degli individui che vivono in questa società.

Nelle mani oggi di questo Governo e domani di un altro? È questo il richiamo che faceva ieri la vice presidente del Senato Emma Bonino, sui numeri che tolgono un

ma l'appello finale è questo: riprendiamo, riguadagniamo spazio per la ragione. Non facciamoci dettare una legge dall'emotività,

Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la discussione su questo argomento ci pone di fronte ad un punto centrale della vita democratica, perché tocca in modo incisivo e per certi aspetti, forse, anche pericoloso la disciplina della libertà della persona. Un antico adagio della vita legislativa, di cui non ricordo la provenienza ma che cito a memoria, dice che i casi difficili producono leggi sbagliate. La storia del caso Englaro lo dimostra. Il fatto sta sotto ai nostri occhi: si propone una legge sul testamento biologico il cui risultato effettivo certo è quello di rendere impossibile il testamento biologico. I promotori, è vero, l'hanno presentato e continuano a presentarlo come un provvedimento che deve riuscire a risolvere un problema di natura universale, però hanno costruito un dispositivo che, al contrario, lo complica ed aggrava. I promotori di questa legge hanno affermato e ripetuto la necessità di colmare un vuoto legislativo. Qui si incontra un primo punto decisivo della questione. Dire che c'è un vuoto legislativo significa infatti poggiarsi su un espediente per sostenere che i giudici che si erano occupati variamente della vicenda Englaro sono stati protagonisti di forzature indebite, hanno creato in modo illegittimo un diritto marginale e hanno invaso l'ambito riservato al solo legislatore.

ha voluto sostenere che la Cassazione, avendo a suo tempo confermato la sentenza della corte d'appello (che permetteva finalmente al padre di Eluana Englaro di avviare alla sua fine naturale la povera figlia), si era così sostituta al potere legislativo. L'accusa era che la Cassazione si era sostituta al potere legislativo e aveva quindi violato il principio fondamentale della separazione dei poteri. Su questa base il Senato ha voluto sollevare un temerario conflitto davanti alla Corte costituzionale ed è stato giustamente bacchettato dalla Suprema Corte. In un certo senso, noi abbiamo esposto il Senato a una figuraccia - viviamo ancora sotto questa aura perché la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto che il Senato ha proposto e, con la massima chiarezza e in pochissimo tempo, che i provvedimenti della magistratura non sono stati usati per esercitare funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere normativo da parte del Parlamento. Ho citato l'ordinanza n. che è inequivocabile. Ciò significa che i giudici avevano agito in piena legittimità. Quando la Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello, essa ha agito nella piena disponibilità dei suoi poteri.

di diritto per sfigurarlo con nuove norme aggiuntive, che, anziché disciplinare l'esercizio di un diritto, di fatto lo impediscono. Dopo l'ordinanza della Corte costituzionale era in realtà dovere del Senato fermarsi. Potevamo e dovevamo fermarci e se proprio pensavamo fosse davvero necessario un sostanziale miglioramento normativo, ci saremmo potuti concedere il tempo necessario per ragionare sul tema e, soprattutto, per ascoltare l'opinione della scienza. Questo è un altro punto fondamentale,

Stiamo parlando di cose che intimamente non conosciamo: noi ragioniamo in termini di diritto, pretendendo di mettere bocca dentro una materia di esclusivo carattere scientifico.

I colleghi della maggioranza hanno voluto misurarsi con il problema scientifico, con esiti penosi, mentre non hanno voluto invece misurarsi con il problema di diritto.

All'improvviso il caso Englaro fa esplodere la necessità della legge. Tuttavia quello che accade in questi giorni dimostra che non si persegue una legislazione necessaria, si cerca una rivincita: questo è quello che sta facendo il Senato, sta cercando la rivincita dello scappellotto preso dalla Corte costituzionale. In quest'Aula abbiamo dovuto ascoltare un'oratoria scomposta, che è arrivata a sostenere che Eluana è stata ammazzata (non dico (non dico da chi, ma è stato detto), e che la decisione legittima che ha posto fine al suo calvario si trasformerà nell'autorizzazione a far morire di fame e di sete i pazienti nella sua condizione: fantasia orribile. Chi usa questo argomento non sa di che cosa parla e affida la capacità di persuasione soltanto alla mistificazione retorica. Basterebbe ascoltare ciò che può spiegare la comunità scientifica, che si occupa per professione delle cure palliative e del trattamento di fine vita, e si vedrebbe allora - a saper ascoltare - che equiparare la rinuncia ad idratazione ed alimentazione artificiali alla negazione di acqua e pane (questo è stato detto, che noi volevamo togliere acqua e pane ad una povera paziente che stava morendo) rappresenta un'autentica falsificazione della realtà. In questa maniera si è giunti all'esasperazione di un conflitto che produce una legge che punta in modo esplicito - è dichiarato, è scritto negli articoli - a limitare il diritto all'autodeterminazione riconosciuto dalla Costituzione.

comma dell'articolo 38, in cui si dice: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio...». Questa è la vita che entra nel testo della Costituzione. Quando poi si parla di inviolabilità, si bara,

Dichiarazione dei diritti dell'uomo, all'articolo 3 si dice che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno dice che la vita è un bene indisponibile. All'articolo 12,

Stabiliamo dunque questo principio assurdo che, in un certo senso, fa riemergere dalla morte filosofica l'idea dello Stato etico, cioè dello Stato che ci dice cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo pensare, come dobbiamo muoverci, perché a questo punto noi stabiliamo che la vita è disponibile per lo Stato. È un'orribile prospettiva

le cure e di morire con dignità - espressione costituzionale - è estremamente chiaro. La decisione della Corte di cassazione, ricordata prima, era ancorata ad una larga serie di norme: ricordo in particolare gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione; la Convenzione su diritti umani la Convenzione su diritti umani e biomedicina del Consiglio d'Europa; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la legge sul Servizio sanitario nazionale del 1978; gli articoli del Codice di deontologia medica,

alle sentenze della Corte costituzionale precedenti. Il criterio di partenza è elementare, vale a dire è il principio del consenso informato da cui deriva il potere della persona di disporre del proprio corpo. Qui sì c'è la disponibilità, ma di disponibilità, vale a dire del potere della persona di disporre del proprio corpo e quindi l'illegittimità di qualsiasi intervento che prescinda dalla sua volontà. Qui incide l'articolo 32 della Costituzione, che vieta qualsiasi trattamento che possa violare il rispetto della persona umana e su ciò si fonda il diritto di rifiutare qualsiasi cura. Il Senato non può prescindere da questo quadro costituzionale. L'intervento del Senato nella legge ha senso solo se consente a ciascuno di esprimere in piena libertà e consapevolezza la propria volontà sulle proprie condizioni di fine vita, nel caso in cui si trovi impedito ad esercitare in quel momento il suo diritto al rifiuto di trattamenti, come hanno potuto fare di recente Welby e Nuvoli. È già successo e dovrà continuare a succedere. Non c'era alcun bisogno di una legge sul testamento biologico. Ma se proprio si deve predisporre una legge sul testamento biologico, allora bisogna che essa sia lineare, chiara e comprensibile, senza sbavature, e affermi con la massima semplicità il diritto di scelta del singolo cittadino. L'articolo 408 del codice civile è chiarissimo: prevede che, in previsione della propria futura incapacità, il cittadino possa designare un amministratore di sostegno affinché siano rispettate le sue indicazioni nel caso in cui si trovi in uno stato vegetativo permanente. Al contrario, la legge qui in discussione vuole proprio impedire il diritto di scelta. Questo è il punto finale. Noi, che difendiamo il diritto di scelta, non vogliamo imporre a nessuno una soluzione che ripugni alla sua coscienza, invece è proprio una grave lesione della democrazia che la maggioranza voglia imporre con una legge a tutti la propria unica soluzione, il prodotto della propria coscienza. Qui compare, lo ricordo ancora una volta, lo Stato che prescrive a tutti i comportamenti che invece dovrebbero essere dettati dalla coscienza individuale. Ma se non bastano questi richiami, che qualcuno potrebbe considerare laicisti, voglio ricordare alle persone di fede chePaolo VI, in una lettera pontificale del 1970 ai medici cattolici, così scriveva: «Il carattere sacro della vita è ciò che impedisce al medico di uccidere e che lo obbliga nello stesso tempo a dedicarsi con tutte le risorse della sua arte a lottare contro la morte. Questo non significa tuttavia obbligarlo a utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza che gli offre una scienza instancabilmente creatrice». Vorrei che fosse apprezzata la potenza semantica dell'espressione del Pontefice «una scienza instancabilmente creatrice», che sposta indefinitamente i confini tra la vita e la morte. Prosegue poi: «In molti casi non sarebbe forse un'inutile tortura imporre la rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabile? In quel caso, il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza, invece di voler prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi condizione, una vita che non è più pienamente umana» - non lo dicono dei laicisti maledetti, lo dice Paolo VI - «e che va naturalmente verso il suo epilogo».

2278: «L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'"accanimento terapeutico". Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha competenza e capacità o, altrimenti, da coloro che ne hanno legittimamente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi del paziente». Questa legge è pessima, è anticostituzionale e probabilmente passerà. Forse sarà cosmeticamente migliorata con l'approvazione di qualche emendamento, ma passerà perché la maggioranza ha la forza per farla passare, però si troverà di fronte un protagonismo civile che non rinuncerà alla sua battaglia. Molti cittadini da poco tempo hanno cominciato a depositare il proprio testamento biologico. La collega Poretti l'ha fatto qui, ma in tutta Italia ci sono ci sono luoghi pubblici in cui si raccoglie il testamento biologico dei cittadini che hanno voglia di farlo. Questa iniziativa avviene senza pubblicità, senza grandi assembramenti, con la massima tranquillità, come si compete all'esercizio del libero

rafforzerà la causa della libertà di scelta nel futuro, sicuramente inevitabile se la legge passerà qui, del rinvio della stessa legge alla Corte costituzionale. Perderemo una votazione e ci appronteremo a sostenere una battaglia civile in tutta la società.

In questi anni la dimensione squisitamente familiare e personale del fine vita si è trasformata in un momento della comunità che, in assenza di regole e soprattutto per l'intervento purtroppo anche un po' prepotente della magistratura,

ha perso la sua naturalezza per divenire oggetto di una legge alla luce della mutata mentalità, di una conseguente consapevolezza della scienza e, permettetemi, di una sproporzione nella visione dell'accettazione dei limiti umani. Di fronte, infatti, al gigantismo dato dalle importanti scoperte scientifiche, ma anche psicologiche e sociali, non accettiamo i limiti della vita, essi appaiono come stridenti di fronte ad un uomo centro della natura, dello spazio e del mondo. Se la scienza medica moderna e lo sviluppo considerevole delle biotecnologie interrogano la vita sia nel momento iniziale sia nel suo evolversi, determinano invece un atteggiamento di paura e di ansia in rapporto alla malattia prolungata, alla condizione di coma, allo stadio precedente la morte e alla perdita di capacità di intendere e di volere. La persona si sente impotente e fatica a discernere tra informazioni contraddittorie e la società e il Parlamento fanno fatica ad assumere delle decisioni. Possiamo dire che il fine vita ci fa paura e ci sentiamo inetti di fronte alle nuove sfide della vita. Esso è vissuto come l'estrema fragilità alla quale non c'è rimedio e si traduce in destabilizzazione. Non voglio citare papi e tanto meno persone autorevoli della Chiesa, voglio citare Platone che, nella sua «Apologia di Socrate», affermava: «Temere la morte, infatti, non è altro, cittadini, che credere di essere sapiente senza esserlo; è credere di sapere ciò che non si sa. Perché nessuno sa se la morte non sia il maggiore di tutti i beni per l'uomo, ma tutti la temono, come se sapessero con certezza che è il maggiore di tutti i mali. Non è ignoranza questa, anzi la più biasimevole, credere di sapere ciò che non si sa? Perciò, davanti ai mali che so essere mali non temerò e non fuggirò mai quelli che non so se siano anche beni». La precarietà della vita ci fa ritenere non degno di essa tutto ciò che se ne discosta o che non assomiglia alla nostra concezione, senza prendere in considerazione che l'uomo è fatto anche di fragilità, come il tempo di attese e di assenze. Voglio ricordare alcuni passaggi dell'Assemblea costituente: lo hanno fatto in molti, ma credo sia doveroso. Ricordo l'articolo 2, l'articolo 13 e l'articolo 32 della Costituzione. La vita è un bene indisponibile della comunità: credo che questo sia un valore in cui ci riconosciamo tutti, anche se poi diamo un'interpretazione applicativa diversa; ritengo, però, che sia un principio importante, prescindendo dalle condizioni cliniche della persona. Altrimenti è come se dicessimo che le persone gravemente disabili non devono essere accompagnate

noi vogliamo realmente difendere la vita, soprattutto nelle sue condizioni di fragilità. C'è poi il benedetto articolo 32, con il secondo comma (lo definisco "benedetto" perché ormai è diventato quello più evocato della Costituzione).

per dire no in modo chiaro ed inequivocabile, come hanno affermato i parlamentari di tutti gli orientamenti politici e culturali. Sono andata a rileggermi il dibattito: lo hanno stabilito per dire no a quelle a quelle sperimentazioni che venivano esercitate su alcune persone e che erano la negazione della dignità umana. Oggi, invece, interpretiamo questo articolo in un modo, non diverso, ma aggiuntivo e dobbiamo tenere conto della diversa interpretazione.

per cui facilmente sconfina nell'autodeterminazione dominante. Mi si opporrà che oggi la scienza ci pone interrogativi inimmaginabili nel 1948, quando è entrata in vigore la nostra Costituzione; la diversa interpretazione è frutto di ricerca, di investimenti e di progressi

la libertà, intesa come possibilità dell'essere umano di scegliere, è la premessa della ricerca della verità. Quest'ultima, però, a livello umano non riuscirà mai ad essere assoluta, piuttosto sarà ricerca del bene possibile. Libertà e verità sono complementari e funzionali l'una all'altra. Se attraverso la scelta si ricerca la verità, è solo con essa che si avrà la libertà. Verità e libertà sono aspetti dinamici che si modificano con la società, o meglio, che si colorano di sfumature diverse secondo i mutamenti sociali e che implicano una responsabilità politica, umana, capace di svincolarsi dalla logica «*valeo ergo sum*», ovvero esisto perché valgo economicamente, che abbia come fine il bene comune. Allora, dobbiamo rifuggire da questo, ma anche da un altro pericolo,

chiedo come sia possibile immaginare uno Stato che impedisca di dire alcuni no. Per poter dire alcuni sì, deve poter dire anche alcuni no! Questa è una legge sicuramente filosofica, nella quale gli Stati moderni, gli Stati della Rivoluzione francese, della «*liberté**, égalité e fraternité*», oggi si riconoscono, ma è anche una legge naturale,

scritto, così, se qualcuno vorrà leggere le mie osservazioni, lo potrà fare. Cosa vogliamo dire con questa legge? In cosa ci vogliamo riconoscere attraverso questa legge? Spero che almeno tutti, tutti, qui dentro, lancino un messaggio positivo, riconoscendosi nella volontà di non abbandonare le persone che vivono questa condizione di fragilità. Mi rivolgo alla maggioranza, e lo faccio con enfasi, e al Governo,

coscienza che non si può riconoscere il principio nei livelli essenziali di assistenza dell'accompagnamento della persona fragile - relatore Calabrò - e poi non prevedere un

che ha dato un segnale importante, perché ha recepito il bisogno dell'accompagnamento del paziente e della sua famiglia, però occorre estendere la platea degli interessati,

rispetto agli stati vegetativi, di aprire uno spazio anche per quei casi di persone che vivono una condizione di perdita di coscienza irreversibile. A questo noi dobbiamo porre attenzione.

delle forme e dell'ampiezza delle dichiarazioni anticipate di trattamento e concerna una visione antropologica cangiante che si scontra e trova la propria inadeguatezza di fronte al confronto con il dolore e l'imperfezione della vita umana. Pensare ogni mattina di dover affrontare il dramma del silenzio di una persona cara, al quale non possiamo dare una tempistica, ci trova arrendevoli e impreparati. Questo è vero. Mette in discussione la nostra stessa esistenza. La legge, allora, deve essere proprio una legge umana, che va incontro a questo bisogno dei familiari. Essere figli del proprio tempo non vuol dire avere una patente di verità assoluta, che anzi costituisce una trappola pericolosa, perché interrompe quella staffetta generazionale che fa ereditare princìpi e valori, il bagaglio fondante di un domani migliore e non di un domani qualsiasi. Vorrei concludere sperando che, così come in Assemblea costituente nomi importanti come Moro, Grassi, Tupini, Tupini, Damiani, Calamandrei, Ghidini, Giua, Nitti, Spallacci, Gullo, che rappresentano tutto l'arco costituzionale di quel tempo e tutte le diverse culture presenti ancora oggi nella nostra società, hanno avuto la capacità di trasmetterci un testo in cui noi oggi ci riconosciamo ancora (è il nostro DNA), anche noi, oggi, migliorando in Aula questo testo, riusciamo a tradurre il bene comune possibile in Non ho quindi né verità né certezze, come credo nessuno in quest'Aula dovrebbe avere, ma sono consapevole della responsabilità delle scelte che stiamo per compiere.

anche dalla cultura politica alla quale fa riferimento o ha fatto riferimento nel corso della sua esperienza, breve o lunga che sia. Vorrei iniziare questo mio intervento dicendo che, per quanto mi riguarda, parto da da quella fase della vita politica del nostro Paese, che colloco nella cosiddetta prima Repubblica, quando sulla scia dell'iniziativa di alcuni parlamentari del tempo, come Loris Fortuna e Antonio Baslini, cominciò

parola, delle cosiddette libertà civili attorno alle quali si registrava in quel tempo un grande distacco fra il senso comune diffuso nel Paese e ciò che invece la società legale e politica rappresentava.

come parte politica e anche come coalizione, che, a partire dalla scorsa legislatura, forse abbiamo avuto l'ambizione di ritenere

e alcuni elementi emersi nella discussione che si è sviluppata attorno a questo tema, segnino questa come una scelta corretta. Siamo andati, secondo me, un po' alla cieca in questa direzione. Infatti, quando sento affermare che la libertà non è un bene assoluto, ma deve sottostare ad un bene collettivo, francamente mi

soprattutto quando questo bene collettivo è stato individuato nei modi e con le forme che ricordo. Quindi, quando sento il relatore che fa questa affermazione così impegnativa, per me ciò è sufficiente per dire che non c'è assolutamente il clima politico, la consapevolezza, l'approccio corretto per discutere di un tema come questo.

sono stati compiuti misfatti terribili. Porto un esempio così forte perché, quando si fa un'affermazione di questo genere, bisogna avere ben chiaro il significato profondo e l'uso che si può fare di certe parole. Per questa ragione, penso che mai come in questa circostanza il bicameralismo perfetto ci aiuterà. Mai come in questa circostanza, quella che abbiamo giudicato una farraginosità del nostro sistema ci sarà forse di aiuto, perché confido molto

tutta la varietà del popolo che mi ha eletto e quindi cerco di esprimere un concetto: dobbiamo stare molto attenti ad evitare di fare una legge applicando la regola del «si fa ma non si dice»,

attorno al quale abbiamo sviluppato discussioni profonde. Sappiamo tutti che cosa c'era dietro quella battaglia civile che abbiamo portato avanti e qual era la filosofia o il punto di vista dominante, prima che quella legge

hanno portato alla nostra attenzione alcuni elementi di riflessione, che mi hanno ulteriormente convinto che non bisogna varare questa legge. Non possiamo discutere fra di noi su questioni come «la vita senza cervello non è vita»,

oppure che «la volontà di non alimentarsi deve essere rispettata solo quando viene espressa in piena lucidità». Ma cosa significa tutto questo? Ciascuno di noi ha fatto delle esperienze di vita dirette. Ho ascoltato l'appassionato ed importante intervento del collega Lusi, stamattina. Io ho vissuto un'esperienza opposta a quella che ha fatto lui,

Ciò che sta dentro la sfera della nostra vita privata e dei nostri affetti non può essere oggetto di una legge. C'è un limite oltre il quale non si può andare, perché - e questo è l'altro punto pericolosissimo non si possono fare mediazioni con i princìpi della Costituzione. I princìpi della Costituzione non sono "anche", come ho sentito dire: sono "prima" di tutto i princìpi della Costituzione, e mi riferisco soprattutto ai princìpi fondamentali. Ognuno di noi poi ha le sue convinzioni etiche e, nella libertà che quei princìpi gli consentono, si comporta come ritiene più opportuno, senza che le sue convinzioni etiche e religiose diventino o possano diventare un vincolo per gli altri. tratta di un punto fondamentale. Diceva bene la vice presidente Bonino nel suo intervento di ieri, che ho molto condiviso: «io non lo farei» non può mai diventare «tu non lo devi fare».

chiudiamo la civiltà politica del Paese che abbiamo faticosamente fatto crescere nel corso di questi anni e paradossalmente, come sento spesso ricordare, anziché cogliere un progresso che si è realizzato nel corso della prima Repubblica nelle battaglie sulle libertà civili e che deve andare oltre, di pari passo con la società che cresce, rischiamo rovinosamente di fare un salto indietro. Ma - concludo su questo - un salto indietro lo facciamo qui, non nella società, qualora dovessimo approvare una legge di questo tipo che secondo me fa a pugni con il buon senso comune.

o agnostici - rispondono nella grande maggioranza dei casi che ognuno deve essere lasciato libero di decidere su questa materia come ritiene più opportuno, il diretto interessato se lo può fare, insieme ai suoi familiari o alle persone a lui più vicine se non non è in grado di farlo. Concludo, signor Presidente, con un auspicio: quello che il bicameralismo perfetto, come ho detto all'inizio, ci sia di grande aiuto

io auspico, tuttavia ci impegneremo in questa direzione), sia l'altro ramo del Parlamento a rappresentare in maniera più opportuna il pensiero libero e democratico di questa nostra Repubblica.

Signor Presidente, Maria, 58 anni, è venuta a mancare cinque giorni fa; e poche settimane prima Angela, Giovanna, Clementina. Quattro donne, quattro lavoratrici tessili, decedute per mesotelioma pleurico negli ultimi mesi, le ultime quattro vittime dell'amianto di un lungo e drammatico elenco che da alcuni anni sta colpendo il paese di Romanengo, in provincia di Cremona. Un paese dove la presenza dell'ex azienda INAR - fabbrica dedita alla tessitura di panni in fibra di asbesto - sta tragicamente segnando la vita di chi lì ha lavorato, in particolare donne. Signor Presidente, oltre ad esprimere la mia solidarietà e vicinanza, convinta di interpretare i sentimenti di tutta l'Aula, alle famiglie colpite dal dramma della perdita dei loro cari così come a coloro che stanno vivendo con angoscia il loro futuro, le chiedo di sollecitare il Governo a dare risposta all'interrogazione a firma mia, del senatore Casson ed altri, con la quale si chiede di rendere operativo il fondo per le vittime dell'amianto, istituito e finanziato con la finanziaria 2008 dal Governo Prodi,

E questo silenzio risulta ancora più amaro e insopportabile, visto che stiamo parlando di uno strumento che non rappresenta solo un sostegno economico, ma che riveste anche una valenza sociale di particolare rilevanza. Chiedo quindi che il Governo dia una risposta urgente su questo tema (risposta già sollecitata in Aula, una settimana fa, dal senatore Casson e che continueremo a sollecitare), affinché alle enunciazioni di circostanza seguano fatti concreti, perché troppi sono i lavoratori che ogni giorno muoiono per essere entrati in contatto con l'amianto. Desidero sollecitare altresì un'accelerazione dei lavori parlamentari di approvazione

Lo dobbiamo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'ex INAR di Romanengo ed alle loro famiglie; lo dobbiamo alle migliaia di lavoratori che ogni anno in Italia muoiono di tumore per esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro. L'enorme debito, morale, civile sociale ed economico che lo Stato hai nei confronti di ognuno di loro, ci impone di non tergiversare oltre, ci impone di mettere questo tema all'ordine del giorno come priorità assoluta e di proseguire con impegno, determinazione e urgenza per chiudere un capitolo drammatico e doloroso nella storia del nostro Paese. *(Applausi tutto il Senato condivide e partecipa alla solidarietà che lei esprime alle famiglie colpite e a quanti vivono (conosco anch'io per esperienza diretta queste situazioni)

risponda all'interrogazione a cui lei faceva riferimento; rivolgerà di nuovo una sollecitazione forte. Per quanto riguarda il disegno di legge che è all'attenzione della Commissione, condivido il suo auspicio. Naturalmente

una parola, a nome mio ed anche del Gruppo del Popolo della Libertà. Sono molto sensibile al tema che la gentile collega Fontana ha sollevato. Due legislature fa (sotto il Governo Berlusconi precedente al Governo Prodi), io, che ebbi l'onore di presiedere la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, come la collega stessa forse ricorda, ebbi ebbi modo di occuparmi, insieme ai colleghi della Commissione, di tale problema. Debbo dire che in quell'occasione furono adottati degli interventi ed anche stanziate delle risorse

ai fondi destinati ad altre finalità, pur importanti, che afferivano al mondo del lavoro. Naturalmente, siccome la coperta generalmente è pregiata ma corta,

esso precedente, e in maniera concreta, anche con interventi economico‑finanziari di non indifferente portata. Vero è, lo dico anche qui senza volere arare il ricco terreno di tale argomento, che le fattispecie sono molto differenziate e anche la giurisprudenza (attivata da molti di noi, anche sul piano professionale, nell'esercizio della professione forense in difesa di molti soggetti danneggiati) si è espressa differentemente, o sul principio dell'effettivo e dimostrato danno,

giuridicamente prioritaria, ma anche non demagogica. Sono certo che, prendendo magari lo spunto dagli atti già depositati dai colleghi sia di maggioranza che di opposizione, si possa in maniera abbastanza paradossale continuare a occuparsi di questa emergenza e intanto apprendere su tutto il territorio nazionale, nelle più varie fattispecie, che abbiamo ancora numerosissime strutture quantità e qualità che con l'amianto continuano ad essere causa di esposizione a rischio di gravi malattie. Mentre cerchiamo di riparare ai danni del fenomeno, questo risulta

nel luglio del 2008, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro, salute e politiche sociali e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

dopo diverso tempo, l'INPS annuncia il riassorbimento di quelle che erano state le erogazioni per equiparare la loro retribuzione,

Grazie,